Presidente, onorevoli colleghi, volevo condividere con voi lo sbigottimento che ho provato ieri nell'ascoltare, all'inizio di seduta, l'intervento del collega Pittella sui tragici fatti che si stanno verificando in Grecia. Uno sbigottimento che mi ha impedito di reagire immediatamente, ma forse questo è stato un bene, visto che, ciò che è ovvio è stato affermato sulla stampa, in particolare su uno dei più prestigiosi e autorevoli quotidiani italiani il «Corriere della sera», da uno dei giornalisti più esenti da quel psicoreato che è il non allineamento al pensiero unico, cioè Federico Fubini. Quello che è successo in Grecia ha una molteplicità di cause, ma è impossibile non menzionarne una, che è il risultato delle politiche di austerità che hanno smantellato, fra l'altro, anche il sistema della protezione civile di quel Paese. I dati sono forniti oggi dal «Corriere della sera»; si parla di tagli di 34 milioni di euro, di un organico dei vigili del fuoco che scende da 12.000 a 8.000 persone e si parla, per le persone che rimangono, di un 79 per cento di vigili del fuoco in sovrappeso e in condizioni di scarsa efficienza fisica perché costretti a ricorrere ad un'alimentazione basata sul *junk food* e, quindi, ovviamente non potendosi permettere un'alimentazione proteica, fuori forma e non fisicamente efficienti.

A me fa piacere che adesso il collega Pittella chieda la solidarietà dell'Europa verso la Grecia, ma quando nel 2012 veniva pubblicato dal Fondo monetario internazionale e imposto a quel Paese un *memorandum*

pari a un terzo di quello che la letteratura scientifica ci forniva, il collega Pittella era vicepresidente vicario del Parlamento europeo; lui era lì

Presidente, molto brevemente e con totale serenità, chiedo al collega che è intervenuto prima di rileggersi tutti gli atti del Parlamento europeo che riguardano la storia della Grexit e il ruolo che ha avuto il Gruppo da me presieduto nel Parlamento europeo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Penso che il ruolo dei socialisti e dei democratici europei sia stato decisivo per salvare la Grecia dalla Grexit, come il primo ministro Tsipras può testimoniare. Quindi non ammetto su questo argomento alcuna lezione da chicchessia.

recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale***

questo decreto-legge arriva in Senato dopo aver assunto alla Camera i contorni di una vicenda preoccupante, a tratti paradossale per come è stata portata avanti dal Governo, dalla maggioranza e dallo stesso ministro Bonafede, che magari avremmo voluto qui in Aula. Sono numerosi gli aspetti che lasciano perplessi, peraltro già da molti sottolineati. Li elenco soltanto giacché non è solo a questi che intendo riferirmi nell'illustrare questa pregiudiziale. Il decreto-legge solleva pesanti interrogativi, tant'è che poche volte si è registrata una così ampia, direi unanime, condivisione di giudizi critici: magistrati, avvocati, amministrativi del tribunale di Bari, tutti ascoltati in Commissione alla Camera e tutti concordi nel contestare aspramente il provvedimento per ragioni, come ho detto, tutte ampiamente evidenziate. Il decreto-legge difetta dei requisiti minimi di necessità ed urgenza, interviene a porre rimedio ad una situazione già mutata (le tende sono già state smontate), intende garantire il regolare svolgimento (lo ripeto: regolare svolgimento!) dei processi e dei procedimenti, ma perviene all'irregolare paralisi degli uni e degli altri, senza aggiungere alcuna soluzione al cambiamento, parola spesse volte usata ed abusata (decreto del cambiamento) senza però che qui, come altrove, si intraveda alcuna reale nuova rotta o novità positiva. rinvia e postula l'individuazione e l'effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti ma patrocinando, in realtà, il disinteresse per tale individuazione, finisce per legittimare una scelta rivelatasi improvvida e a dir poco inopportuna, così come evidenziato da molti organi di informazione. poi, violandola, sulla ragionevole durata del processo garantita dall'articolo 111 della Costituzione e produce certamente ed inevitabilmente ritardi sui tempi necessari per far ripartire i processi: due mesi di sospensione hanno la capacità, autorevolmente evidenziata, di produrre più di qualche anno di ritardo. Moltiplica incredibilmente gli adempimenti necessari per quelle notifiche a tutte le parti processuali, stimate in un numero non inferiore a 60.000, che invece la soluzione delle tende, per quanto mortificante, aveva tentato di evitare e risolvere. Colpisce princìpi di garanzia fra i quali quello del *favor rei*, impermeabile espressione di retroattività di condizioni di sfavore. Differenzia indebitamente posizioni processuali omologhe, esponendo gli indagati o imputati di Bari a posizioni processuali di svantaggio rispetto ad altri indagati in altre parti d'Italia, in scoperta violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Potrei proseguire a lungo, seguendo la scia delle critiche alle quali, invece, faccio rinvio per ragioni di sintesi e di sensatezza dialettica. Aggiungo solo due ulteriori notazioni che aggravano la sensazione di irragionevolezza del decreto-legge e confortano l'invito ad arrestarne l'approvazione. Il decreto-legge non solo si lascia giudicare incostituzionale, inutile, paradossale, ma aggiunge difetti di economicità, annunciandosi costoso e certamente irrispettoso della clausola di invarianza finanziaria, la quale non potrà essere rispettata nei fatti. Al di là del ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e a una citazione per danni del Ministero della giustizia dinanzi al giudice di pace di Bari, con annessa eccezione di legittimità costituzionale, il rischio è di alimentare un risultato deflattivo per le aspettative economiche che si legano al regolare e puntuale esercizio della giurisdizione, in questo caso penale. Valgono per tutte le aspettative di ragionevole durata, ivi comprese quelle di giovani avvocati su cui, ingiustamente, graveranno i costi economici legati alla paralisi della loro attività professionale. In aggiunta, la sospensione del corso della prescrizione viene fatta applicare «del tutto irragionevolmente, anche a quei reati che, oltre ad esser stati commessi anteriormente, hanno visto i relativi processi essere rinviati ben prima della sua entrata in vigore, ed a data successiva ai termini del 30 settembre 2018 da esso fissati». Indifferenti alla condizione di emergenza verrebbero tuttavia attratti in una disciplina eccezionale, alla quale avrebbero potuto benissimo rimanere estranei. Il che lascia immaginare profili di incostituzionalità che saranno certamente eccepiti alla ripresa del procedimento. Signor Presidente, questa nostra pregiudiziale non è dunque pretestuosa, ma ha il senso di un richiamo a condizioni di equilibrio e buon senso, che rendono auspicabile, da parte del ministro Bonafede, un doveroso ripensamento e una correzione di rotta, senza dubbio coraggiosa, ma necessaria - mi verrebbe da dire - tipica di quel senno del poi che non esprime debolezza ma, al contrario, dimostra quella intelligenza che dovrebbe guidare i nostri pensieri

*(FI-BP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, che vedo seguire molto attentamente questo dibattito sulla pregiudiziale costituzionale, credo che sia necessario fare una premessa. Dobbiamo metterci d'accordo se il rispetto della Costituzione debba essere uguale per tutti e valere per sempre o se, invece, il rispetto della Costituzione abbia prospettive prospettive differenti a seconda della posizione che si assume in Parlamento. Dico meglio: nella scorsa legislatura un partito, che oggi è maggioranza e ha responsabilità di Governo, ha fatto del rispetto della Costituzione la propria bandiera, il proprio cavallo cavallo di battaglia. Oggi, vedo che la posizione assunta da questo partito è diametralmente opposta a quella sostenuta nella scorsa legislatura. *(Applausi che avessimo due posizioni diverse e cioè il rispetto della Costituzione da parte della opposizione e invece il non rispetto della Costituzione da parte della maggioranza, perché questo sarebbe veramente un fatto gravissimo che andrebbe censurato in tutte le sedi. in tutte le sedi. Signor Presidente, mi rivolgo a lei, perché vedo che è l'unica che segue con attenzione questo dibattito. Sentiamo parlare e leggiamo sui giornali che il ministro Bonafede (che avremmo avuto avremmo avuto il piacere di avere in Aula per poter interloquire, perché siamo anche disponibili, possibilmente, a cambiare idea se qualcuno ce ne dà una ragione o ci dà una spiegazione) ha fatto della funzione dell'ascolto un suo elemento di riconoscimento: il ministro Bonafede ascolta, il ministro Bonafede partecipa. l'ascolto fine a se stesso, che non tiene conto dei suggerimenti, delle proposte, delle iniziative, è assolutamente inutile ed è una presa in giro per questo Parlamento. *(Applausi dal Gruppo signor Presidente, che questo decreto-legge sia un antipasto rispetto a quello che dovremmo aspettarci nel corso della legislatura. Non vorrei nemmeno che fosse parte del progetto di realizzazione di quel principio e di quella filosofia - che abbiamo letto sui giornali - che appartiene alla Casaleggio associati, che addirittura pronostica l'inutilità del Parlamento, quasi che l'elezione da parte dei cittadini a suffragio universale sia mortificata e sostituita

sia stata tenuta in considerazione, quasi che fosse stato già deciso che il decreto-legge doveva essere approvato così com'era e del dibattito e del confronto con quelle organizzazioni che saranno chiamate ad adempiere non importava non importava niente a nessuno. È vero, questo Governo non ha alcuna responsabilità rispetto alla situazione drammatica che si è creata presso gli uffici giudiziari del distretto di Bari, ma questo non autorizza il Governo a emanare un provvedimento strampalato, inutile, dannoso e incostituzionale. Mi rivolgo ai colleghi della Lega, ai quali chiedo di non lasciare che la giustizia sia un campo esclusivamente destinato al MoVimento 5 Stelle; la responsabilità di Governo è collettiva: la Lega può e deve intervenire anche nel settore della giustizia, perché il provvedimento ha molteplici aspetti incostituzionali. Innanzi tutto, non vi sono i presupposti di urgenza; lo abbiamo sentito, ma non lo diciamo noi. Lo hanno detto i parlamentari della maggioranza nel dibattito alla Camera e lo hanno detto

mentre relativamente al terremoto dell'Aquila c'è stata una dichiarazione di emergenza, qui si è voluto emanare un decreto-legge senza alcuno stato di emergenza; il che, quindi, non giustifica il decreto-legge.

3 vieta la disparità di trattamento: qui siamo in presenza di una disparità di trattamento *ratione loci*, e cioè, il cittadino che ha la disavventura di trovarsi nel distretto di Bari ha un trattamento diverso da tutti gli altri cittadini del Paese. Questo non è possibile. Abbiamo la lesione dell'articolo 111 della Costituzione: la ragionevole durata del processo. Colleghi, la sospensione della prescrizione, che sembrerebbe un rimedio per affrontare una situazione emergenziale, non fa altro che favorire la prescrizione dei processi. Lo ha detto il presidente del tribunale di Bari: poter ripristinare la situazione con questo decreto-legge porterà via dieci anni. In dieci anni si prescriveranno migliaia di processi, con tanti ringraziamenti da parte della criminalità e con tante proteste di migliaia di parti lese, che sono violentate da questo provvedimento.

ma come è possibile andare a modificare l'istituto della prescrizione con effetto retroattivo, quando tutti sappiamo - ce l'hanno insegnato all'università, ma ce l'ha ricordato la Corte costituzionale con ben tre sentenze, nel 2006, nel 2008 e nel 2014 - che l'istituto della prescrizione

il principio della buona fede ai nostri interlocutori e abbiamo sempre la speranza che in qualunque momento vi possano essere atti di resipiscenza e mi auguro che ci sia, in questa circostanza, un momento di resipiscenza. Invito il Governo a volersi a volersi fermare per evitare una brutta figura, per evitare ancora una volta la sanzione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, alla quale si è rivolta l'avvocatura barese con fondamento, con legittimità e con coerenza e del magistrato civile, di fronte a quale è stato citato il Ministro della giustizia per risarcimento dei danni. In definitiva, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, noi riteniamo che manchino la situazione di urgenza che legittimerebbe la sospensione dei processi e la possibilità di entrare a piedi uniti sul principio della irretroattività della norma penale, per non parlare di tutte le altre violazioni di carattere di merito che ci sono e delle quali discuteremo in prosieguo ove questa pregiudiziale dovesse essere respinta. Abbiate un attimo di riflessione ed evitate di portare avanti questo provvedimento, che creerà danni enormi alla giustizia barese già malata per conto suo.

come emerge dalle questioni pregiudiziali che ci accingiamo a votare, il testo in esame produce alcune perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale. In particolare, nel decreto-legge non sembra che ricorrano quei presupposti di necessità e urgenza che la Costituzione, all'articolo 77, pone chiaramente come indispensabili per il legittimo utilizzo della decretazione d'urgenza. È vero che abbiamo rappresentato l'urgenza di risolvere i problemi del tribunale di Bari, ma questa urgenza doveva essere applicata alla ricerca di una soluzione, individuando un edificio che potesse ospitare stabilmente il tribunale e tutti i suoi uffici. Questa della sospensione dei termini è una misura decisamente drastica, che è stata adottata in passato in casi assolutamente estremi, come in occasione di gravi calamità naturali, che rendevano di fatto impossibile la prosecuzione ordinaria della giurisdizione. Erano quindi disposizioni realmente urgenti, volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione presso i tribunali. È grave che il decreto-legge non sia stato adottato conseguentemente ad una dichiarazione di uno stato di emergenza, e che le disposizioni siano state di fatto determinate da una negligenza nella gestione della macchina giudiziaria di Bari. È grave il fatto che il Ministro, nell'adottare tale provvedimento, si sia concentrato soltanto sulla sospensione dei termini dei procedimenti non abbia contestualmente individuato la disponibilità di una sede pubblica idonea per trasferirvi gli uffici del tribunale di Bari e della procura. Una soluzione logistica era ciò che si attendeva, questo sì con urgenza. Questa drasticità rischia di ledere diritti costituzionalmente garantiti, che sono stati già ampiamente illustrati nei precedenti interventi. Vorrei però soffermarmi sull'articolo 24 della Costituzione, che sancisce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e statuisce che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. inoltre l'articolo 111 della Costituzione, che stabilisce che la giurisdizione è attuata mediante il giusto processo e dispone che la legge assicuri la ragionevole durata del processo. pregiudiziali viene rilevato quanto emerso nel corso delle audizioni svoltesi durante l'*iter* parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento: la procura della Repubblica di Bari ha sottolineato, in particolare, che l'adozione del decreto-legge non è affatto priva di oneri. Viene correttamente osservato che le cancellerie si troveranno costrette a predisporre almeno 60.000 notifiche, al fine di convocare le nuove udienze, senza considerare i costi inutilmente sostenuti per consulenze e intercettazioni: tutte attività che vengono messe nel nulla e sono relative a processi, che non arriveranno certamente a conclusione. La stima di 60.000 notifiche determinerà anche un allungamento dei processi e un costo - il Ministero parla già di una *task force*, che dovrà essere poi impegnata alla ripresa dell'attività - e segna anche un allungamento dei termini di prescrizione, con conseguenze opposte in relazione agli obiettivi che si spera si intendano perseguire. Quindi, concludendo, le disposizioni del decreto-legge in esame presentano evidenti profili di incostituzionalità, con particolare riguardo agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, posto che si tratta di una sospensione dei termini, ovvero di una evidente lesione del principio di legalità. Inoltre il decreto-legge in esame si riferisce a procedimenti penali pendenti, senza specificare a quale data gli stessi procedimenti debbano risultare tali. Per questo motivo abbiamo presentato un emendamento, al fine di fare chiarezza sul punto, perché anche l'indeterminatezza, di questi tempi, genera perplessità

Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò ora esclusivamente sulla pregiudiziale di costituzionalità; nel caso in cui

alla legge e la certezza della pena, in relazione alla considerazione, ormai consacrata dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui il decorso della prescrizione non è un termine processuale, ma un principio sostanziale. La Corte costituzionale si è espressa tante volte nel definire la prescrizione un elemento della punibilità.

il Parlamento a maggioranza decidesse che invece il provvedimento è costituzionale, ci riserviamo di entrare anche nel merito per annunziare la nostra opposizione.

Si è arrivati al punto che il 12 luglio il ministro Bonafede è dovuto correre in fretta e furia in Aula alla Camera per cercare, tra le altre cose, di spiegare perché fosse stato soltanto un giornale a fare gli accertamenti necessari e dovuti che il Governo avrebbe dovuto fare in maniera del tutto autonoma a tempo debito. Vorrei ricordare a tal proposito che se non fosse stato per le richieste del Partito Democratico e delle altre opposizioni il ministro Bonafede quel giorno non sarebbe andato molto oltre qualche *post* o qualche *tweet*. Ciò per dire innanzitutto quanto il Governo tenga in considerazione il ruolo del Parlamento. Lo vorrei ricordare senza polemica: il Governo sbaglia a offendersi se il Parlamento pone dei problemi su un provvedimento che, tramite un decreto-legge, sospende i termini di un processo penale. Lo ripeto: tramite un decreto-legge sospende i termini di un processo penale. Si tratta, come è evidente, di una scelta a dir poco abnorme. Non può offendersi allora il Governo se dalle opposizioni viene un'offerta di aiuto per togliersi, con ogni evidenza, da una situazione di palese difficoltà in cui lo stesso Governo è andato a infilarsi. Non può valere la difesa del Parlamento quando si è opposizione e il suo svilimento quando si diventa maggioranza. Invece è quello che, ahimè, abbiamo visto accadere fino ad oggi, fino a questo momento. Per ciò innanzitutto chiediamo al Governo un atteggiamento diverso nel considerare i problemi oggettivi che il decreto-legge pone. Non lo dico io, non lo sostiene solo il Partito Democratico; ve lo hanno detto, quasi a voce unanime, magistrati, avvocati e amministrativi del tribunale di Bari ascoltati in Commissione alla Camera. Dovete spiegare a loro perché sono stati chiamati in audizione e poi di tutti i loro suggerimenti puntuali e mirati non si è fatto assolutamente nulla I nostri dubbi sul decreto-legge erano forti in partenza e con il passare dei giorni - ahimè! - si sono rafforzati, signor Presidente. Si è deciso di agire tramite decreto-legge rinvenendo la necessità e l'urgenza di un provvedimento di sospensione. Lo abbiamo detto: a noi preoccupa che il Ministro lo abbia rivendicato più volte, sostenendo che, di fronte a una situazione definita drammatica, l'obiettivo è togliere le tende. Ha detto bene il mio collega Stefano. E questo - ahimè - lo ha ripetuto anche il Ministro in Parlamento, purtroppo. Noi, insomma, stiamo votando un decreto-legge per togliere le tende che la Protezione civile ha nei fatti già smontato in una giornata, e, quindi, senza cambiare di una sola virgola la situazione di Bari. E allora vorrei capire dove stanno l'urgenza e le sue ragioni oggettive; quelle ragioni che due sentenze della Corte costituzionale richiamano come prerequisito necessario per poter utilizzare uno strumento normativo come questo. Parliamo di misure urgenti e indifferibili che dovrebbero garantire il regolare svolgimento dei processi e dei procedimenti: così è scritto già nella rubrica. Peccato che nel decreto-legge non esista alcun intervento che vada nel senso di questa garanzia. La verità è un'altra, anche se il Ministro della giustizia la nega insistendo nel dire che nel decreto-legge non rientra l'individuazione del nuovo immobile. È sufficiente invece leggere la relazione tecnica al decreto, anche se forse questo Governo è allergico alle relazioni tecniche *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lì c'è scritto che la sospensione fino al 30 settembre rappresenta «il periodo necessario a consentire che l'amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per l'individuazione e per l'effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti». Quindi è lo stesso Governo che parla dell'immobile come parte essenziale per risolvere il problema. Vedete, allora, che il problema c'è. c'è. Ad oggi non c'è alcuna certezza che in un tempo breve venga scelto un immobile adeguato, a meno di perseverare nell'errore compiuto dal Ministro individuando un edificio che, già solo per le dimensioni, è palesemente inadatto a ospitare il palazzo di giustizia, come del resto ha detto il presidente delle camere penali. E questa è solo una delle criticità che emergono dalla scelta compiuta e - almeno a quanto apprendiamo dalle dichiarazioni del Ministro - al momento sospesa. Ricordo a tutti che alla Camera il Ministro ha dichiarato che avrebbe fatto le verifiche necessarie. Ma di queste verifiche ad oggi - sono passati diversi giorni - non c'è alcuna traccia. riguarda i modi e i tempi con cui l'intera procedura dell'individuazione dell'immobile è stata condotta dal Governo. Il Parlamento ha saputo - lo dicevo all'inizio del mio intervento - solo dagli organi di stampa che la nuova sede era stata acquistata pochi mesi fa, dopo tanti anni di abbandono, da un fondo pubblico per conto di una società il cui socio di maggioranza risulta essere un imprenditore - possiamo dirlo - alquanto spregiudicato, quantomeno per relazioni e investimenti. Noi del Partito Democratico al garantismo non facciamo deroghe, neanche in questa vicenda. Ma la fretta è pessima consigliera. Ed è più che lecito, anzi direi doveroso, non solo per il PD ma per tutti noi, sollevare dubbi sull'opportunità di procedere con tanta celerità e solerzia per poi arrivare a una decisione che non solo nei fatti è molto costosa per lo Stato, ma in sostanza non è nemmeno risolutiva del problema edilizio che coinvolge il tribunale di Bari. Direi che i dubbi sono più che leciti. Rendiamoci conto che, arrivati al 30 settembre, il rischio che in questo contesto si rendano necessari altri allungamenti e ulteriori proroghe c'è e al momento è davvero alto; un rischio tanto concreto che il rappresentante del Governo in Commissione giustizia, la scorsa settimana, non lo ha potuto negare. Ha però preferito rinviare la risposta a non si sa quando; d'altra parte, è coerente con le generiche e fumose affermazioni e precisazioni date dallo stesso Ministro. Allora gli esponenti del Governo e della maggioranza farebbero bene a fermarsi fino a che sono ancora in tempo, prima, cioè, di andare avanti e trovarsi tra qualche mese nella situazione di essere costretti ad assumersi quelle responsabilità che oggi invece il Ministro della giustizia rifiuta di prendersi. Noi pertanto ribadiamo ancora una volta quanto abbiamo già ripetuto a gran voce in questi giorni: il Ministro acconsenta all'attribuzione di poteri straordinari per sé o per chi intende delegare, in modo da avere la facoltà di individuare e rendere operativo un immobile realmente adatto a ospitare la sede del tribunale di Bari. C'è poi un altro punto, che non è di poco conto e ci preoccupa forse ancora di più: la ragionevole durata del processo, garantita dall'articolo 111 della nostra bella Costituzione. Mi sarò distratta, ma non ricordo che la deroga a questo principio fosse contenuta nel vostro contratto di Governo. Forse era addirittura troppo anche per voi. La sospensione provocherà ritardi sui tempi necessari per far ripartire i processi. Tutto questo, nei prossimi anni, sarà di grave inciampo per il regolare svolgimento della funzione giudiziaria. Altro che misura per l'efficienza della giustizia! È tutto il contrario e lo ha ripetuto il Presidente del tribunale di Bari: se sospendete le attività per due mesi, fate un danno che sarà recuperabile soltanto in dieci anni. Ben dieci anni, signor Presidente! Inoltre, questo provvedimento tocca in maniera sconsiderata l'istituto della prescrizione. Vuol dire entrare a gamba tesa sulla irretroattività della legge penale, ma significa soprattutto impedire per un tempo indefinito il regolare svolgimento della giustizia penale, il risultato - e non è un risultato di poco conto - che un indagato, per il solo fatto di essere parte di un procedimento incardinato a Bari, si troverà in una posizione processuale di svantaggio rispetto ad altri indagati in altre parti d'Italia.

si rischia di avvicinarla, dato che si stimano in almeno 60.000 le notifiche che dovranno essere ripetute, dalla citazione in giudizio, alla data, all'avviso dei testimoni. Stiamo creando un pericolosissimo precedente, senza neanche - ahimè - avere chiaro quale sia lo scopo del decreto-legge. Quando questi problemi sono stati posti da tutte le forze politiche e dagli operatori, da parte del Governo c'è stato completo silenzio, direi un assordante silenzio. Finora non è stato ascoltato neppure il Comitato per la legislazione, che chiedeva di circoscrivere il perimetro dei procedimenti coinvolti, indicando almeno a quale data si dovesse considerare la pendenza, come è stato fatto per il decreto sospensivo dopo il terremoto del 2016. Ditemi voi, allora, a cosa serve dire di ascoltare, se poi degli avvertimenti e dei suggerimenti ricevuti non se ne fa assolutamente nulla? Tutto questo peraltro non è a costo zero per nessuno: non lo è per le parti coinvolte nel processo, perché state toccando i diritti dell'imputato e dell'indagato, ma anche quelli delle persone che hanno subito l'offesa; non lo è per l'efficienza della giustizia, perché il regolare esercizio della giustizia penale subirà un grave colpo, per i magistrati e per gli avvocati. In una settimana sono arrivati già un ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e una citazione per danni del Ministero della Giustizia. Temo che ne arriveranno altri. Anche su questo sarebbe bastato ascoltare. Nessun beneficio poi avranno i cittadini, che vedranno colpita la loro giusta la loro giusta aspettativa. Non è ancora a costo zero per le casse dello Stato: trovo grave che non siano state indicate le cifre di copertura. Concludo, signor Presidente: queste sono le motivazioni che stanno dietro alla nostra questione pregiudiziale. Il Governo aveva la possibilità di dimostrare nei fatti di voler rendere più efficiente il nostro sistema giustizia. Ha perso un'altra occasione. Noi gli chiediamo, con la nostra questione pregiudiziale, di fermarsi, perché sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Signor Presidente, illustri rappresentanti del nostro Governo, gentili senatrici, gentili senatori, partiamo da una situazione oggettiva: l'immobile, destinato a suo tempo in via provvisoria a palazzo di giustizia di Bari, è diventato, grazie all'inerzia di tutte le autorità coinvolte, definitivamente provvisorio. Già nel 2012 - e il Governo non era della Lega e non era del MoVimento 5 Stelle - intervennero modifiche strutturali di consolidamento. A maggio di quest'anno, a seguito di una perizia chiesta dall'INAIL, che sanciva il pericolo di crollo asintomatico - cioè da un momento all'altro - della struttura, il Comune di Bari si è visto costretto a revocare l'agibilità. Curioso che venga imputato al ministro Bonafede, l'unico Ministro della giustizia che si sia attivato per il problema, il fatto di essersi attivato. Non ci sarebbero necessità e urgenza. Abbiamo una situazione in cui i lavori dei procedimenti penali e civili si svolgono in una tendopoli, in condizioni che, ben lungi dall'essere di pace processuale, rasentano i termini della Convenzione i termini della Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra. Ma qui qualcuno fa eccezione di costituzionalità. Ma quale costituzionalità, quando abbiamo termini di sospensione dei procedimenti, che sono termini di sospensione non della sola prescrizione, ma anche dei termini di difesa - a proposito di lungaggine dei processi - di tre mesi. I suggerimenti dei colleghi del PD e della senatrice Valente sono sempre ben accetti, qualora costruttivi. Peccato però che negli ultimi anni ai vostri Governi non abbiate saputo dare i giusti suggerimenti, considerata la situazione della

La vostra risposta al sovraffollamento delle carceri è stato un decreto svuota carceri, travestito da riforma dell'ordinamento penitenziario.

Presidente, il Governo del cambiamento è già cominciato e continuerà.

di un'emergenza che perdura da anni, nell'inerzia di chi aveva la responsabilità non di lanciare suggerimenti, ma di fare. Oggi viene criticato un Ministro che adotta un provvedimento di urgenza, perché - ripeto - svolgere dei processi in una

Di conseguenza, noi riteniamo che le proposte di questione pregiudiziale siano assolutamente infondate. E per quanto riguarda la proposta di questione pregiudiziale presentata dal Partito Democratico, aggiungo una valutazione di assoluta vergogna. È vergognoso. Sono stati al Governo! È vergognoso!

Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, intendo tener fede a un codice di condotta che mi sono dato fin dal giorno in cui l'Esecutivo ha chiesto la fiducia di quest'Assemblea. Una condotta, cioè, di opposizione rigorosa ma mai pregiudiziale e tantomeno strumentale. Starò dunque ben attento a distinguere i cascami di inadeguatezze strutturali che affliggono l'apparato pubblico del nostro Paese (fra questi, l'onta di una situazione ampiamente nota come insostenibile, eppure trascinata negli anni) da inadeguatezze nuove ma a mio avviso non meno gravi. E se del passato non si può dare colpa a un Governo in carica da poche settimane, del presente non si vede a chi altro bisognerebbe chieder conto.

Proprio ieri, preparando questo intervento, ho ritrovato una documentazione risalente al 2010 nella quale il problema della sede di via Nazariantz veniva già definito "annoso" (e in effetti andava avanti da molto). In quell'occasione il piano terra del palazzo di giustizia era stato invaso dalla fuoriuscita di liquami dal sistema fognario: efficace metafora di una situazione lasciata colpevolmente a imputridirsi. Per lunghi anni ci si è chiesti come si potesse tollerare che gli uffici preposti al controllo di legalità venissero lasciati in un edificio fuori legge. Per lunghi anni abbiamo tutti ascoltato, e alcuni di noi supportato, gli accorati appelli degli operatori della giustizia del capoluogo pugliese. Per lunghi anni ci siamo scontrati con le ottusità di quanti hanno ostacolato, per ragioni che speriamo fossero solo ideologiche, soluzioni strutturali e innovative che pure erano a portata di mano. Il risultato è che magistrati, avvocati, cancellieri, parti civili e imputati si sono trovati per la prima volta accomunati nel ruolo di vittime. Ma era questa la soluzione da adottare o piuttosto questo decreto non rappresenta, per restare in tema, una pena accessoria? Dapprima si è passati da un'inerzia quasi ventennale ad una reazione dettata da una sorta di isteria; dal «tutto va bene, madama la marchesa» a operazioni improvvisate, disordinate e precipitose, quasi che si fosse nell'imminenza di un crollo. E così si è finiti a celebrare processi in una tendopoli. Poi, maneggiando con sconcertante disinvoltura un istituto come la prescrizione - che, come hanno detto meglio di me i colleghi Vitali e Stancanelli, l'orientamento della giurisprudenza giurisprudenza costituzionale qualifica come istituto di diritto penale sostanziale, assoggettato al principio di legalità - si è stabilito che a pagare il prezzo dell'inerzia del passato e delle isterie del presente fossero i cittadini. Con picchi di notevole amenità, come ad esempio una sospensione dei termini che opera anche nel mese di agosto, quando notoriamente di processi non se ne celebrano. E senza che nel frattempo ci si sia preoccupati di mettere in campo misure straordinarie per far fronte a un *surplus* di adempimenti che, solo a voler menzionare le notifiche da rinnovare, la procura della Repubblica di Bari ha quantificato nel numero di 60.000. Forse - lo dico ai colleghi del Governo - rispetto al rischio che tanti processi vadano in fumo, questo problema è leggermente più significativo del decorrere dei termini a ferragosto. La prescrizione, dicevamo, non è un orpello procedurale; probabilmente il ministro Bonafede la considera un fastidioso ostacolo, se non proprio un agente criminogeno, ma in realtà è un istituto di civiltà che comporta la rinuncia dello Stato alla potestà punitiva per ragioni legate al trascorrere del tempo, quando questo trascorrere del tempo è determinato dalla stessa amministrazione della giustizia. Non è un caso che il nostro ordinamento colleghi la sospensione dei termini del processo alle richieste di rinvio da parte dell'imputato. È invece inaudito che a fermare il decorrere della prescrizione, addirittura per processi non ancora iniziati, sia l'incapacità dello Stato e delle sue articolazioni di garantire l'esercizio della giustizia in in un luogo idoneo, e ciò per ragioni non imprevedibili, come ad esempio un terremoto, ma talmente prevedibili da essere note da quasi un ventennio. se questo decreto è il biglietto da visita delle iniziative di Governo in tema di giustizia, l'esordio è decisamente una stecca. Vedete, signori del Governo, io non credo che la politica possa essere misurata solo in termini di consenso immediato presso la platea di riferimento del proprio agire. Ma, quando in un ambito così divisivo come quello della giustizia penale si riesce nel miracolo di mettere d'accordo in un colpo solo avvocati e magistrati, e si suscitano pesanti critiche tanto sulla gestione procedimentale dell'emergenza quanto sulle soluzioni edilizie prospettate per tamponarla in via provvisoria, forse, al posto vostro, qualche domanda me la porrei. Non si tratta di rinverdire il vecchio adagio dei «tanti nemici, tanto onore»; qui non ci sono nemici, ci sono soltanto cittadini che rischiano di pagare due volte per mancanze altrui. Astraendoci per un attimo dalla stretta attualità, e assumendo il caso Bari a emblema di disfunzioni antiche e strutturali, sarebbe opportuno che questa vicenda rappresentasse

è proprio il caso di dirlo - grande come una casa. E questo problema riguarda le sedi giudiziarie non meno che le scuole e gli altri edifici di importanza strategica, in quanto adibiti a servizi pubblici essenziali. Quand'anche il tema della supervisione tecnica e manutenzione del patrimonio immobiliare fosse da considerare soltanto in termini di spesa, comunque si tratterebbe di una spesa doverosa perché afferisce alla sicurezza dei cittadini e, come abbiamo visto a Bari, alla continuità nell'erogazione dei servizi. Ma il punto è che monitorare in via sistematica, manutenere, consolidare, mettere in sicurezza gli edifici che ospitano le nostre scuole, i nostri tribunali, i nostri ospedali, consentirebbe addirittura di realizzare un risparmio, economie di scala a beneficio dei conti pubblici. Spesso infatti ci si interroga sull'ammontare della spesa corrente per la supervisione e la manutenzione edilizia; troppo raramente ci si chiede quanto costi gestire le emergenze che non si è preparati ad affrontare. Peraltro - consentitemi un inciso la situazione nella quale si trovano le province, per quel che riguarda scuole e strade, sta fortissimamente peggiorando la situazione. Come vedete, colleghi del Governo, non siamo inclini a fare di tutta l'erba un fascio. Sappiamo bene che ci sono problemi atavici e problemi che invece ineriscono al presente. in premessa, questa vicenda richiama responsabilità antiche e responsabilità nuove. Quelle antiche non le dimentichiamo. Su quelle nuove siamo chiamati oggi a pronunciarci in quest'Aula, senza pregiudizi ma con la fermezza di un giudizio che nel merito è profondamente negativo e, per quel riguarda questo decreto, non cadrà in prescrizione.

chi solleva questa pregiudiziale dice una cosa vera, ma anche una cosa infondata. Quella vera e condivisibile è che, in effetti, la situazione del tribunale di Bari era nota fin dal 2012, o addirittura dal 2010,

quindi recentissima, ha reso evidente che il tribunale di Bari non poteva più essere utilizzato per il rischio di crolli senza preavviso. Quindi a maggio 2018 è intervenuto un *factum principis*, e cioè un'ordinanza del Comune di Bari che ha revocato l'agibilità. Risulta, inoltre, che ad agosto verrà addirittura emesso un ordine di sgombero. Pertanto, è soltanto da maggio 2018 che questo tribunale, per lungo tempo oggetto dell'incuria delle precedenti amministrazioni, è divenuto non più agibile. Siffatta situazione quindi, di recente emersione dal punto di vista dell'inagibilità,

la Corte costituzionale dice che i casi straordinari di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 lasciano un largo margine di elasticità e il Governo può decidere di provvedere con decreti d'urgenza, citando alcuni casi: in casi cioè di eventi naturali, comportamenti umani e anche provvedimenti di poteri pubblici. Quindi, c'è una assimilazione di questi fatti che rende evidente come nel caso specifico si sia agito né più né meno che come si è agito in passato. Aggiungo - e qui vengo alla seconda eccezione che viene che sempre il Governo, quando ha sospeso i termini dei processi e dei procedimenti, ha anche agito sulla sospensione della prescrizione e mai, in tutti i casi che vi ho citato in precedenza, la Corte costituzionale è intervenuta a censurare il fatto. Peraltro, nei casi in cui per legge vengono sospesi i processi e procedimenti si debba o si possa incidere anche sui tempi di prescrizione, sospendendola, è un principio immanente del nostro sistema, che è stato anche cristallizzato nell'articolo 159 del codice penale. non esiste una questione costituzionale sul punto. Mi limito, peraltro, a dire che la sospensione è soltanto di tre mesi, interviene in un caso analogo a quelli precedenti e consente a questo Governo di fare, appunto in pochi mesi, quello che i precedenti Governi non hanno fatto in due legislature.

per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici

Signori senatori, la notizia della scomparsa di Sergio Marchionne, le cui drammatiche condizioni di salute erano da giorni note, non può non trovare in quest'Aula un momento di ricordo e di riflessione. Non è oggettivamente questa la sede per una valutazione approfondita sul suo operato e sugli obiettivi manageriali raggiunti. Sono certa che su questo nei prossimi anni sarà inevitabile una dettagliata analisi storica. Ciò che in questo momento desidero sottolineare è il tratto umano e l'indiscussa italianità di un grande professionista che ha saputo portare il prodotto italiano nel mondo; un percorso non isolato che rimanda ai pionieri dell'imprenditoria italiana che hanno contribuito a fare grande il nome dell'Italia nei mercati internazionali. Tutti coloro che hanno conosciuto Sergio Marchionne sono rimasti inevitabilmente colpiti dal legame che ha sempre mantenuto con la sua terra d'origine, l'Abruzzo, con le radici profonde della sua famiglia; una famiglia che ha conosciuto il dramma dell'esodo istriano-dalmata e che poi, attraversando l'Atlantico, ha cercato e trovato quel riscatto comune a tanti figli della nostra Patria. Per quanto riguarda gli aspetti industriali, il mio auspicio è che i frutti delle sue scelte e delle sue intuizioni non vengano dispersi, ma possano continuare a vivere per il bene di FCA, dei lavoratori italiani e di tutto il Paese. Ai parenti e alla famiglia Agnelli Elkann desidero esprimere i sensi del mio profondo cordoglio per la perdita di un professionista illuminato, un caro amico e un padre straordinario. Invito quindi tutti i colleghi ad osservare un minuto di raccoglimento.

*relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge che andiamo ad esaminare riguarda la conversione in legge del decreto-legge n. 84 2018, finalizzato a incrementare per l'anno 2018 la capacità operativa sia della Guardia costiera del Ministero della difesa sia degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libico, libico, attraverso la cessione a titolo gratuito di unità navali italiane, nonché la fornitura delle risorse necessarie alla manutenzione di questi mezzi e lo svolgimento di specifiche attività addestrative e di formazione per il personale libico. Ricordo innanzitutto che le questioni della messa a disposizione di unità navali italiane alla Libia, della loro manutenzione e dello svolgimento di mirate attività addestrative non sono nuove, essendo state oggetto di accordi bilaterali e di cooperazione tra i nostri due Paesi fin dal 2009, nel quadro delle attività volte al controllo e alla sicurezza dei mari, nonché al contrasto dell'immigrazione irregolare e del traffico di esseri umani. Gli accordi bilaterali sottoscritti in passato hanno portato anche all'adozione di specifici protocolli tecnico-operativi riguardanti anche le attività addestrative. Ricordo soprattutto il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008. Tale Trattato riaffermava l'impegno delle parti ad operare per il rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilità, in particolare nella regione del Mediterraneo, e definiva un nuovo partenariato bilaterale, prevedendo (all'articolo 19) l'intensificazione della collaborazione bilaterale nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina, nonché la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche da affidare a società italiane. Ricordo inoltre che alla Dichiarazione di Tripoli del gennaio 2012, con cui l'Italia ha assicurato il proprio sostegno politico al processo di pacificazione nazionale in atto in Libia, ha da ultimo fatto seguito anche il Memorandum d'intesa sottoscritto nel febbraio 2017, che stabilisce l'impegno reciproco dei due Governi a completare il sistema di controllo dei confini del sud della Libia previsto dal Trattato del 2008. Il provvedimento che andiamo ad esaminare si pone, dunque, in stretta continuità con l'impegno italiano degli ultimi anni, indirizzato al rafforzamento degli strumenti operativi a disposizione di Tripoli per esercitare la sua autorità nel controllo delle acque antistanti la costa libica, puntando al rafforzamento degli accordi di collaborazione sottoscritti nel recente passato. Del decreto-legge evidenzio in primo luogo i requisiti di straordinarietà e di urgenza, stante - mi sembra ovvia - la necessità di contribuire in tempi brevissimi al consolidamento delle capacità operative della Libia, conformemente alle richieste del Governo di Tripoli, nell'attività di controllo e vigilanza delle proprie acque territoriali, anche al fine di garantire la sicurezza della navigazione nel Mediterraneo e di porre un argine all'immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani che si muovono dall'Africa verso l'Europa e che da troppi anni stanno interessando proprio la rotta del Mediterraneo centrale. Per il nostro Paese, in particolare, il rafforzamento della collaborazione bilaterale con la Libia costituisce un elemento di estrema rilevanza, non solo per continuare a perseguire l'obiettivo del contenimento della pressione migratoria, che proprio dalle coste libiche quasi sempre si origina, ma anche per una tutela più adeguata delle stesse frontiere esterne, italiane e dell'Unione europea, oltre che per un'azione efficace di contrasto alla criminalità organizzata internazionale e di prevenzione dai potenziali rischi di infiltrazione di soggetti contigui alle organizzazioni terroristiche. Andando ai contenuti del provvedimento, evidenzio che il disegno di legge di conversione si compone di un solo articolo che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2018 a far data dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge, a sua volta, si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente: in ordine alle cessioni di unità navali alla Libia

4). Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge dispone, per le singole componenti delle Forze armate e di polizia, la specifica autorizzazione alla cessione, a titolo gratuito, di dodici unità navali, nonché alla relativa autorizzazione di spesa. È previsto in particolare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze siano autorizzati alla cessione a titolo gratuito di dieci unità navali CP, classe 500, fra quelle in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e di due unità navali da 27 metri, classe Corrubia, fra quelle in dotazione alla Guardia di finanza. Tale cessione avviene conformemente a specifiche intese con autorità libiche e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni internazionali ed europee in materia di sanzioni internazionali. Per il ripristino in efficienza e il trasferimento delle unità navali dall'Italia alla Libia è autorizzata una spesa complessiva, per il solo anno 2018, di 1,15 milioni di euro. L'articolo 2 del decreto-legge in esame stabilisce, a sua volta, l'autorizzazione a una spesa complessiva di 1,37 milioni di euro, fino al 31 dicembre 2018, per la manutenzione delle singole unità navali cedute e lo svolgimento di attività addestrative e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. Pertanto, gli oneri complessivi del provvedimento sono quantificati in 2,52 milioni di euro per il solo anno 2018, alla cui copertura l'articolo 3 provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Allo scopo, si utilizzeranno accantonamenti relativi ai Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il prospetto degli oneri, come potete facilmente vedere dai documenti allegati, è dettagliato nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame.

mentre, a nostro giudizio, esprime tutta la sua valenza e portata, soprattutto in considerazione della strategia che il Governo vuole e vorrà attuare in merito alla gestione del fenomeno migratorio. di un tema sul quale ci confrontiamo e alle volte ci scontriamo anche con durezza, che ogni giorno tocca il nostro popolo, soprattutto le fasce più deboli della nostra popolazione. Quindi, è un tema che non possiamo affrontare con superficialità, ma che ci deve vedere tutti coinvolti nell'interesse comune della nostra Nazione. Ebbene, a questo proposito, partendo dalla posizione di Fratelli d'Italia, noi da sempre siamo favorevoli alla collaborazione con i Paesi del Nord Africa nel controllo del flusso migratorio. A ciò risponde, evidentemente, il contenuto del decreto-legge I rapporti con questi Paesi - con la Libia, in particolare - vanno quindi sicuramente incrementati. Ricordo a noi tutti come già dal 2007-2008 (quindi con un Governo di centrodestra)

Noi aggiungiamo che la questione dell'Africa e delle migrazioni va affrontata da parte di tutti, anche nella consapevolezza che

Nello specifico, per quanto riguarda il provvedimento in sé, Fratelli d'Italia ha fatto già rilevare i problemi contenuti nel decreto-legge quando è arrivato in Commissione e, in particolare, in Commissione affari Ha fatto rilevare che il decreto si presentava piuttosto scarno e monco in alcune parti; addirittura vi erano problemi di copertura, vi era l'assenza assoluta di chiarimento della relativa diminuzione del capitale del patrimonio dello Stato perché, cedendo un bene dello Stato, il suo patrimonio va diminuendo e non era previsto nulla in termini numerici al riguardo nel decreto giunto in Commissione.

Fortunatamente, grazie anche all'intervento di Fratelli d'Italia in Commissione affari esteri, il Governo ha risposto su questi tre aspetti, dando una caratterizzazione finalmente

che riguarda la salvaguardia della capacità operativa; stiamo cioè trattando di una cessione a titolo gratuito di motovedette, di barche e di navi alla Libia, per controllare e pattugliare le coste. Siamo tutti d'accordo: ben venga. Però, nel far questo, andiamo a togliere questi mezzi navali alla Guardia costiera e alla Guardia di finanza. Noi, allora, abbiamo chiesto in sede di Commissione affari esteri, ma anche in sede di Commissione finanze, rassicurazioni al Governo circa il fatto che il venir meno delle motovedette non inficiasse la disponibilità strutturale delle nostre Forze

Concludo ringraziando per l'attenzione e sperando che il Governo abbia davvero a cuore il fenomeno delle politiche migratorie, ma abbia anche a cuore che le nostre strutture territoriali non vengano meno negli strumenti che ci servono per pattugliare e difendere le nostre coste.

Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi presenti in quest'Aula, sono particolarmente onorato di poter intervenire per la prima volta in questa Assemblea e lo sono ancora di più per la rilevanza del decreto in esame. Come è a tutti noto, l'Italia sta vivendo in questo periodo e ormai da anni una situazione particolarmente critica con riguardo ai fenomeni migratori che stanno interessando l'intero Paese. Risulta pertanto necessario intervenire con provvedimenti e con accordi che mirino a facilitare il ripristino del controllo di tali flussi, proseguendo nella direzione che in più occasioni l'attuale Governo fin dal suo insediamento ha delineato e mostrato di voler seguire. Il decreto-legge che oggi discutiamo persegue il duplice obiettivo di voler limitare l'ormai insostenibile traffico di esseri umani nel Mediterraneo, insostenibile in termini economici ma ancor più in termini di costi umanitari. Basti pensare, a tal proposito, alle migliaia di persone che, con la speranza di trovare migliori condizioni di vita, lasciano il proprio Paese d'origine e non riescono spesso a raggiungere le coste di alcun Paese europeo, perdendo nel peggiore dei casi la propria vita.

che il decreto-legge in esame prevede, ha l'obiettivo di voler finalmente intervenire a favore di un'auspicata e ormai più che necessaria gestione corretta dei flussi migratori, con particolare interesse a quelli provenienti dalla Libia, attribuendo massima rilevanza all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani e alla salvaguardia della vita umana in mare. Va, a mio avviso, interpretata allo stesso modo la fornitura delle risorse necessarie alla manutenzione di tali mezzi e lo svolgimento di specifiche attività addestrative e di formazione per il personale libico. Tali provvedimenti non sono nuovi e rientrano pienamente nel sentiero tracciato da numerosi e rilevanti accordi intercorsi tra i due Paesi negli ultimi dieci anni. Come ricordato da più colleghi in sede di Commissione, tale decreto prosegue, infatti, quanto già intrapreso dal 2009, anno a partire dal quale, con una serie di accordi bilaterali tra Italia e Libia, si è deciso, agendo con fine di cooperazione, di intervenire per contrastare l'immigrazione incontrollata e il traffico di esseri umani e per garantire in termini di sicurezza la navigazione del Mediterraneo centrale, il tratto di mare più battuto e interessato dai flussi migratori. Con il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista, firmato a Bengasi a Bengasi il 30 agosto 2008, si sono infatti mossi i primi passi in questo senso, manifestando la volontà di porre rimedio, tra le altre cose, proprio all'immigrazione clandestina. La collaborazione tra i due Paesi in tale direzione ha visto, infatti, la promozione di pattugliamenti congiunti delle coste libiche tramite la cessione di motovedette italiane alla Libia già a partire dal 2007, le cui proroghe hanno visto similmente nel 2010 la cessione di quattro unità navali dal Governo italiano al Governo libico. Superata la guerra civile libica, dopo che, tra l'altro, le appena citate unità navali sono rimaste danneggiate, nell'epoca successiva alla morte di Gheddafi, si è proseguito sulla linea della cooperazione e sul rafforzamento del rapporto di amicizia tra Italia e Libia e nel 2012, con la Dichiarazione di Tripoli, il Governo italiano, nella persona del presidente Monti, ha nuovamente sancito la volontà di voler supportare con azioni congiunte e con il proprio sostegno politico il processo di pacificazione interno al Paese. Proseguendo, è con il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato di Libia e la Repubblica italiana, firmato dal presidente del Consiglio presidenziale Fayez al-Sarraj e dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni Silveri a Roma il 2 febbraio 2017, che si è voluto proseguire su questa linea sancendo il comune impegno alla stabilizzazione del Paese e al Governo dei flussi di migranti clandestini e di contrasto ai traffici illeciti. Questo breve *excursus* storico, che mi ha visto citare brevemente i punti salienti del rapporto di cooperazione e partenariato che contraddistingue a partire dal 2009 le relazioni tra Italia e Libia, si rende necessario per evidenziare che la conversione del decreto-legge, oggi all'esame dell'Assemblea, ha lo scopo di proseguire nella stessa direzione che i Governi che ci hanno preceduto, seppur in situazioni diverse e con minor vigore, hanno tracciato. Le finalità di tale decreto sussistono, infatti, nel voler fornire ulteriori strumenti per contenere gli ormai incontrollabili flussi migratori, anche in un'ottica di tutela delle frontiere esterne e di prevenzione di potenziali rischi di entrata nel nostro Paese di persone vicine o facenti direttamente parte di organizzazioni terroristiche che potrebbero minare la sicurezza del nostro Paese. Se si vuole perseguire tale obiettivo, che vede la cooperazione come un elemento cardine ed imprescindibile per la risoluzione e il governo dei flussi migratori, non più gestibili per l'Italia, un tale decreto risulta, di fatto, non solo necessario ma d'obbligo. L'attuale flotta a disposizione della guardia costiera libica non risulta in alcun modo sufficiente a garantire un controllo adeguato delle frontiere né un adeguato soccorso nei frequenti casi di necessità, tristemente registrati sempre più frequentemente e che questo Governo vuole assolutamente impedire. Le quattro motovedette cedute dall'Italia e, precisamente, dal Governo Berlusconi e quindi da quello Gentiloni Silveri sono state dismesse. Le dieci imbarcazioni classe 500 che verranno con tale accordo cedute alla Libia, della lunghezza di dieci metri ed in vetroresina, così come le due unità navali classe Corrubia di 27 metri e capaci di raggiungere i 43 nodi e dall'autonomia, a velocità di crociera di 21 nodi, di 800 miglia rappresentano sicuramente dei mezzi necessari per agire con efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale provvedimento risulta, poi, ancor più giusto e degno di apprezzamento se si considera che l'Italia andrà così a coadiuvare con un importante contributo il controllo di un confine marittimo che non è solamente italiano ma europeo.

il decreto-legge di cui si dispone la conversione, persegue l'esigenza di incrementare la capacità operativa delle autorità costiere libiche mediante la cessione, a titolo gratuito, di dieci unità navali in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e due in dotazione alla Guardia di finanza, da destinare alle attività di controllo e di sicurezza per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani, e alle attività di soccorso e di salvaguardia della vita umana in mare. La complessità delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio e la necessità di contenerne la pressione, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, anche in un'ottica di tutela delle frontiere esterne e di prevenzione di potenziali rischi di infiltrazioni da parte di soggetti contigui alle organizzazioni terroristiche, hanno indotto il Governo ad adottare il presente provvedimento in condizioni di urgenza. La Libia costituisce ormai da anni il principale porto di partenza dei flussi migratori che attraverso il Mediterraneo tentano di raggiungere l'Italia e l'Europa. Da quando il regime del dittatore Muammar Gheddafi è stato rovesciato, ovvero dall'ottobre 2011, il Paese nordafricano non è mai riuscito a compiere una transizione democratica. I trafficanti di esseri umani approfittano di tale situazione di instabilità politica ed economica, con il risultato che i migranti sono vittima di abusi continui. Il provvedimento si inserisce nell'ambito dei vigenti accordi bilaterali e di cooperazione tra Italia e Libia: Trattato di Bengasi, Dichiarazione di Tripoli e specialmente il Memorandum d'intesa del 2 febbraio 2017, che, tra gli altri punti, stabiliva il rafforzamento della sicurezza alle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana. Questa intesa ha consentito di mettere a disposizione della guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici motovedette italiane, nonché di provvedere alle attività di manutenzione e di addestramento del personale. Da parte sua, l'Unione europea addestra gli ufficiali della guardia costiera libica sin dall'ottobre 2016 nell'ambito dell'operazione Sophia, lanciata nel luglio 2015 con lo scopo di contrastare l'attività illegale dei trafficanti di esseri umani lungo il Mediterraneo centrale. Ad oggi, sono 188 gli ufficiali libici che hanno completato la formazione. Ne è conseguito che, a partire dal luglio 2017, gli sbarchi in Italia sono progressivamente diminuiti, tanto che, dal 1° gennaio al 24 maggio 2018, sono giunti sulle coste italiane 10.808 migranti, di cui 7.103 provenienti dalla Libia. Si tratta di una diminuzione di quasi il 78 per cento rispetto ai dati dello stesso periodo del 2017. Inoltre, nei primi tre mesi del 2018, la guardia costiera libica ha compiuto più di 4.100 operazioni di salvataggio in mare nella tratta del Mediterraneo centrale, tra la Libia e l'Italia, raggiungendo una cifra pari a quasi il doppio rispetto ai 2.500 soccorsi effettuati dalle navi delle ONG nello stesso periodo. È quindi indispensabile dare un seguito a misure che si sono rivelate estremamente utili. In attesa che la componente manutentiva libica acquisisca le necessarie competenze per garantire il funzionamento delle dodici unità navali da trasferire, il decreto-legge prevede la fornitura di un supporto logistico fino al 31 dicembre 2018. È prioritario garantire adeguati *standard* di sicurezza della navigazione nel Mar Mediterraneo, al fine di gestire correttamente le dinamiche dei fenomeni migratori, specialmente di quelli provenienti dalla Libia, che vedono l'Italia da anni in prima linea. Fra il 2014 e il 2017, ovvero nei quattro anni in cui è stato più attivo il flusso dal Nord Africa, sono arrivate via mare in Italia ben 623.000 persone, per cui il nostro Paese possiede senz'altro un *know-how* sulle attività di soccorso in mare che deve essere necessariamente trasmesso ad altri per una fruttifera collaborazione allo scopo di contrastare in modo veramente efficace il fenomeno. Questa non è una misura da considerarsi risolutiva, ma è soltanto un contributo, un supporto a una visione più complessa e globale che questo Governo sta garantendo con il proprio lavoro, con determinazione e alacremente.

all'interno di una sostanziale strategia di continuità con quanto fatto dai Governi precedenti, finalizzata a portare stabilità al Paese. il relatore, così come i due colleghi che mi hanno preceduto, hanno fatto in parte la cronistoria dei rapporti bilaterali tra Italia e Libia, a partire dal Trattato di amicizia del 2008, che era orientato e rafforzare i legami tra i due Paesi, per arrivare al Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato di Libia e la Repubblica italiana, firmato a Roma, dal Presidente

il provvedimento di cui stiamo discutendo oggi nel rafforzare il nostro supporto tecnico direttamente nelle acque territoriali libiche, al fine di contrastare efficacemente il traffico illecito di esseri umani, tuttavia con la cessione delle unità navali e il rafforzamento della Guardia costiera libica si affronta solo la parte finale di un problema molto più complesso del fenomeno migratorio in atto nel Mediterraneo centrale. Tra l'altro - come accennava anche il relatore - c'è una forte preoccupazione che deriva dal rischio sul fronte della minaccia terroristica, perché

c'è una sorta di diaspora che rischia di incrociare i flussi migratori. Quindi certamente c'è un potenziale rischio di infiltrazione, perché chi fugge cerca la strada più

vanno bene le cessioni navali ma, nello stesso tempo, credo che tutti siamo consapevoli che una crisi complessa come quella legata ai flussi migratori possa venire affrontata solo con una strategia multidimensionale, che non può non comprendere anche un quadro di accordi in ambito europeo e con i Paesi di origine dei flussi, come è stato detto. La possibilità di rimpatriare un maggior numero di immigrati regolari, si scontra sempre con la riottosità dei Paesi di provenienza e il problema - diciamocelo - è un po' sempre quello. Tornando al Memorandum del 2017, è il caso di sottolineare le molteplici attività e iniziative attuate nelle fasi finali dei Governi precedenti nella direzione di un maggior controllo dei flussi.

quindi la cessione delle navi, ma non va abbandonata la rete realizzata, ad esempio, con i sindaci delle città della Libia più coinvolte dal traffico degli esseri umani con le tribù (i cosiddetti guardiani del deserto). Dobbiamo quindi sostenere, anche finanziariamente e comunque in generale, tutte quelle regioni colpite dal fenomeno dell'emigrazione. Occorre anche tenere ben presenti gli accordi che sono stati fatti sul confine subsahariano in Libia, quindi con i Paesi del Ciad, del Mali e del Niger, al fine di rafforzare la capacità di controllo dei confini marittimi e terrestri di quei Paesi, coinvolgendo anche l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (INM) e l'UNHCR, che svolgono un ruolo molto importante

In questo senso, va richiamata la necessità di migliorare gli *standard* di visibilità dei centri di permanenza in Libia, dove vengono accolti questi disperati che attraversano il deserto. Sempre in questo contesto - voglio ricordarlo

Poi vi sono, ancora, tutti gli accordi di riammissione con i Paesi a forte vocazione migratoria. Alcune intese sono già state fatte,

dalla capacità di tessere relazioni internazionali ed è quindi necessario un approccio meno improntato ai gesti esemplari, oltretutto fatti sulla pelle delle persone, secondo noi poco efficaci efficaci a lungo termine, perché l'immigrazione, come penso sappiamo tutti, è un fenomeno strutturale e non può essere gestito attraverso politiche emergenziali.

sui media, in particolare negli ultimi mesi. È un problema serio e siamo consapevoli che, sotto la superficie di questa grande crisi, il problema risieda nelle gravi instabilità che costellano il contesto odierno e nello stato delle relazioni internazionali. Non la faccio lunga, ma è comunque essenziale ragionare su quale sia la risposta più adeguata. La realtà ci dice che le crisi di oggi richiedono capacità irraggiungibili per un singolo Stato e, di conseguenza, un approccio che sia almeno almeno verosimile non può prescindere dall'operare in ambito multilaterale e dal costruire una strategia politica prima che operativa.

il provvedimento si inserisce in un contesto che condividiamo, seppure va richiamata, come dicevo, la necessità di implementare e di rafforzare altre importanti funzioni fondamentali, che sono alla base

ossia di rendere esplicita la volontà, la collaborazione e l'onestà dell'Italia nei confronti di un mondo che soffre e chiede aiuto e nei confronti dell'Europa stessa. Il nostro Governo ha scritto nel contratto che nei tavoli dei negoziati europei avrebbe ricoperto un ruolo da protagonista, con l'intento di far rispettare i diritti e i doveri dell'Unione europea e lo stiamo facendo. Il carattere deciso, caparbio e irremovibile del nostro Ministro dell'interno ci sta garantendo rispetto e un'improvvisa collaborazione da parte di Stati europei che fino a ieri erano miopi al problema. Abbiamo infatti riaperto una coscienza egoisticamente chiusa, affinché ci sia una equa e responsabile ripartizione del ricollocamento dei richiedenti asilo. Solo grazie alla nostra leale forza politica e morale siamo oggi ascoltati, considerati e rispettati. La boriosità e il menefreghismo anch'esso egoisticamente assunto da alcuni *leader* europei sono oggi rimandati al mittente. In modo leale, forse anche duro per alcuni, il nostro *leader* Matteo Salvini ha interpretato la volontà degli italiani, ovvero quella di offrire amore ai popoli che soffrono, ma pretendendo impegno comune, regole comuni e risposte serie e veloci. Questa strategia organizzativa fa seguito al Trattato di Bengasi del 2008, al quale riconosciamo la lungimiranza di chi vedeva allora nella Libia un *partner* per cooperare in accordi bilaterali che determinano lotta al terrorismo e alla criminalità, lotta al traffico illecito, soprattutto di stupefacenti, e all'immigrazione clandestina, nonché un alleato sulle sponde nordafricane, fornitore di energia, gas e petrolio. Apprezziamo la continuità strategica, anche se di debole efficacia sui tavoli europei, del precedente Governo; abbiate perciò anche voi dell'opposizione il coraggio e la correttezza di apprezzare di apprezzare il lavoro del nostro Esecutivo e il ruolo assunto nei confronti di un'Europa che scaricava sull'Italia tutte le responsabilità economiche, politiche, legali, umanitarie e sociali e che si nascondeva egoisticamente dietro patti, trattati e accordi firmati, con la consapevolezza degli enormi svantaggi arrecati. Penso poi al ruolo assunto nei confronti di organizzazioni private autoproclamatesi legittime e autoreferenziali, organizzazioni senza alcun obbligo di pubblicità di bilancio e che non svelano con trasparenza finanziatori e finalità. un Governo che ha il merito di lavorare per renderci un sentimento che purtroppo da troppo tempo manca, cioè quello di Patria; una Patria che in Europa conti e si faccia sentire. Rivendichiamo pertanto orgogliosamente la volontà di cedere a titolo gratuito ben dodici unità navali siamo orgogliosi di fornire altresì supporto, addestramento ed istruzione operativa, di fornire sacrificio di uomini e donne italiani, formazione e copertura finanziaria per una spesa complessiva di 1,15 milioni di euro. Diamo un segno tangibile aggiungendo dodici unità operative alle quattro motovedette della Libia vecchie e limitate. Per salvare davvero le vite umane e combattere davvero i trafficanti di morte occorre operare un contrasto già nei luoghi di partenza, perché lì è la cupola e perché impedire ad uno scafo insicuro di partire significa evitare tragedie in mare. Noi in Italia accogliamo volentieri e senza trattati i rifugiati veri; deve finire il *business* delle cooperative dell'accoglienza indegna e ricca di lucro. Oggi aiutiamo le istituzioni libiche, non solo con soldi ma con mezzi, formazione, uomini e tecnologie avanzate che consentiranno di reprimere efficacemente la malvagità dei trafficanti impuniti. Questo provvedimento ci costa anche la consapevolezza di sacrificare le dodici unità, sfilandole ad altri impegni del nostro territorio, ma la fame di umanità e di pace ci rende forti, fieri e fiduciosi. Chiediamo di non strumentalizzare la colpevolezza e di non augurarsi qualche tragedia per poter alzare in modo ipocrita il dito e dire «lo avevo detto». C'è poco da dire, infatti, sulla nostra onestà e lealtà. Il nostro Governo non lascerà mai morire le persone e renderà onore alle vittime del mare, punendo il sistema degli infami traghettatori di morte e di chi ha guadagnato soldi sporchi di sangue.

il decreto-legge n. 84, licenziato il 2 luglio scorso, prevede la cessione da parte dell'Italia alla Libia di dodici navi da destinare alla sicurezza della navigazione nel Mediterraneo; una cessione a titolo gratuito di motovedette in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto, alla Guardia costiera e alla Guardia di finanza, per garantire in particolare la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità, in primo luogo, all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani e, in secondo luogo, immediatamente dopo, alla salvaguardia della vita umana in mare. Sono previsti i fondi necessari a garantire la manutenzione delle unità e lo svolgimento di attività addestrative e formative del personale libico; c'è uno stanziamento totale di circa 2,5 milioni di euro attraverso fondi che sono in riserva dei Ministeri interessati. Va ricordato che già in passato si è provveduto ad accordi che prevedevano sostegni di questo tipo da parte del nostro Paese alla Libia. In data 29 dicembre 2007 era stato siglato un protocollo per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, accompagnato da un protocollo tecnico-operativo siglato che prevedeva un pattugliamento congiunto con la cessione in uso di motovedette motovedette e attività di addestramento, formazione, assistenza e manutenzione dei mezzi. Ad esso è seguito, poi, un protocollo aggiuntivo tecnico-operativo, siglato il 29 dicembre 2009. I periodici decreti-legge di proroga delle missioni internazionali hanno autorizzato, a partire dal disegno di legge n. 8 del 2008, la partecipazione del personale della Guardia di finanza italiana alle missioni bilaterali in Libia di supporto alla Guardia costiera libica e la spesa per

4 unità navali. Tali unità sono rimaste danneggiate nel corso della guerra civile libica e sono state riportate nuovamente in Italia per essere riparate, dopodiché sono state custodite dal Corpo della Guardia di Finanza nel comprensorio di Miseno per essere poi riconsegnate alla Libia nell'aprile

unicamente verso porti libici, ma la Libia oggi, purtroppo, non può offrire ancora, secondo la normativa, un porto di sbarco cosiddetto sicuro. Anche i più recenti rapporti delle Nazioni Unite e i giudici di Ragusa e Palermo nelle loro sentenze escludono, alle attuali condizioni, che la Libia possa offrire porti sicuri di sbarco, tenuto conto anche della precaria situazione politica e della mancata sottoscrizione libica della Convenzione di Ginevra sui rifugiati. In tal senso, appare quanto mai urgente, quindi, un impegno dell'Italia a favorire la stabilizzazione e la normalizzazione politica del Paese. Nel maggio 2009 - dobbiamo ricordarlo - l'allora Governo italiano, che aveva messo in esecuzione i citati accordi, fu condannato dalla Corte d'Europa dei diritti dell'uomo (sentenza 23 febbraio 2012) per respingimenti considerati illegittimi, eseguiti dalla Guardia di Finanza verso Tripoli, in quanto - si legge nella sentenza - costituivano violazione dell'articolo 3 (tortura e trattamento inumano) della Convenzione europea dei diritti umani, perché la Libia non offriva alcuna garanzia di trattamento secondo gli *standard* internazionali dei richiedenti asilo e dei rifugiati e li esponeva ad un rimpatrio forzato.

La sentenza fu quindi una completa smentita delle giustificazioni addotte a suo tempo dall'Italia a sostegno della pratica del respingimento in acque internazionali dei profughi e migranti clandestini provenienti dall'Africa settentrionale. A oggi, purtroppo, la Guardia costiera libica non ha i mezzi e gli assetti organizzativi per salvaguardare effettivamente la vita umana in mare. La sua capacità di ricerca e salvataggio è molto al di sotto degli *standard* internazionali imposti dalle convenzioni e dal regolamento (IMO). Il supporto, in termini di mezzi e addestramento, che il Governo italiano offre oggi alla Guardia costiera libica non basterà a cambiare questa realtà e a fornire un'effettiva garanzia sulle capacità di soccorso della Guardia libica dall'oggi al domani. Così come il mero riconoscimento di una zona SAR libica non comporta, di per sé, la qualifica automatica di porto sicuro, senza dimenticare le difficoltà di aprire *hotspot* nei Paesi del Sahel, sul piano sia politico, che umanitario. È inutile nascondersi la difficoltà e la complessità di un problema non facile risoluzione, ma che necessariamente il Governo italiano dovrà affrontare con coraggio, tempo e pazienza. Migliorare l'operato della Guardia costiera libica è solo un piccolo passo di un lungo cammino.

sostiene l'obiettivo del Governo italiano di aiutare e rafforzare il contrasto al traffico di esseri umani e ai barconi della morte che partono dalle coste libiche e attraversano il Mediterraneo. Quindi, noi siamo favorevoli agli aiuti che il decreto-legge in esame offre alla Libia, in esecuzione, tra l'altro, di accordi già presi anche da precedenti Governi. Certo, la situazione è molto complicata e la crisi è molto complessa, per cui riteniamo che l'unica vera soluzione sia quella del blocco navale. Per impedire le morti nel Mediterraneo, bisogna impedire ai barconi della morte di partire. Questo è, secondo noi, l'unico modo per porre fine, finalmente, a questa tragedia. Come del resto fece il Governo Prodi nel 1997 e nel 1998 nei confronti dell'Albania. Questo, però, cari colleghi, non deve significare sguarnire la Guardia costiera italiana di mezzi importanti e fondamentali per i compiti che le nostre Capitanerie di porto stanno assolvendo già

a sostituire quanto prima i mezzi che sono stati sottratti alla nostra Guardia costiera. Si tratta di mezzi importanti e fondamentali perché - lo voglio ricordare, colleghi - tre motovedette vengono sottratte alla Puglia e due alla Sicilia e queste motovedette, così come le altre, svolgono un ruolo fondamentale nella salvaguardia dei nostri confini. modo, voglio ricordare a tutti i colleghi che nella Provincia da cui provengo c'è Goro, la più grande marineria dell'Adriatico per numero di imbarcazioni immatricolate (circa 1.300), dove l'unica motovedetta disponibile è stata sottratta per essere mandata in Libia.

Ho letto la risposta di alcuni esponenti della Lega sulla stampa locale, i quali hanno affermato che, quanto all'unica motovedetta che è stata sottratta alla nostra Guardia

perché il Governo aveva già deciso di fornire di modernissime motovedette le Capitanerie alle quali venivano sottratte queste dieci (più due) imbarcazioni. Ebbene, la realtà purtroppo è un'altra, perché il Governo ha respinto l'emendamento di Adolfo Urso, in base al quale questo impegno sarebbe stato scritto nero su bianco: oggi abbiamo soltanto delle promesse, ma le promesse non ci bastano. La realtà è ben diversa. La realtà è che la Capitaneria di Goro, come altre Capitanerie, ad oggi sono già più di trenta giorni che non ha alcun mezzo navale per effettuare il soccorso in mare e per contrastare le attività illecite che deve contrastare. Buon senso vorrebbe che prima di sostituire e di mandare via un mezzo - definito obsoleto mentre in realtà non è così, perché il mezzo era efficientissimo ed è stato mandato in cantiere solo per cancellare le scritte e i numeri identificativi della Guardia costiera prima e non dopo, si desse l'alternativa per garantire l'efficienza e la funzionalità della nostra Guardia costiera. Quindi noi siamo d'accordo in linea di principio, ma non siamo d'accordo nel metodo, perché, ripeto, non si può sguarnire in questo modo i già precari strumenti a disposizione della nostra Guardia costiera e delle nostre Capitanerie. a nome di Fratelli d'Italia, il relatore e il Governo a riflettere sull'emendamento che abbiamo proposto ed esprimere parere favorevole alla sua approvazione.

Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, colleghi senatrici e senatori, il decreto-legge oggi in esame, già trattato in Commissione esteri, è una misura necessaria per dare seguito all'operato del Governo e del Ministro dell'interno in materia di gestione dei flussi migratori, oggetto degli accordi bilaterali sottoscritti in passato con manchevole risultato. La cessione gratuita di motovedette alla Libia si propone l'obiettivo di rafforzare la cooperazione Grazie a questo decreto-legge anche la Libia potrà contribuire ad un soccorso in mare che sia più efficace e che sia volto a prevenire possibili naufragi nel Mar Mediterraneo. La salvaguardia di vite umane deve sempre essere al primo posto di qualsiasi azione politica. infatti consapevoli che la politica non si fonda su sensazioni o prime impressioni, ma sul realismo e cioè quella capacità di leggere e interpretare le situazioni reali per arrivare ad una soluzione di qualità, quella soluzione, realismo e capacità che sta dimostrando oggi l'attuale Governo e la sua maggioranza, grazie agli interventi mirati decisi dal ministro dell'interno, Matteo Salvini. Non solo: la cooperazione con il Governo libico porterà anche a disincentivare i viaggi nel Mar Mediterraneo e, di conseguenza, anche la tratta degli esseri umani nel Nord Africa e quindi i viaggi dei migranti che partono dell'Africa subsahariana e dal Corno d'Africa, restituendo e rispettando infine la dignità umana. Voglio inoltre sottolineare come questo decreto-legge vada nella direzione di responsabilizzare anche la Libia. È un aiuto che è al tempo stesso un atto dovuto per un obiettivo comune: i canali illegali che favoriscono la tratta degli esseri umani devono essere chiusi definitivamente. L-SP)*. Non possiamo assolutamente accettare che questi rischiosi viaggi della morte siano consentiti. È inaccettabile che un rifugiato politico, già perseguitato nel proprio Paese d'origine, debba rischiare la vita per ottenere una protezione che è un suo diritto, come abbiamo sempre sostenuto. A tal fine sarà necessario consentire ai veri rifugiati la possibilità di usufruire di un canale legale che tuteli la loro sicurezza e che consenta un'analisi anticipata o almeno un primo filtro della domanda d'asilo, già prima dell'utilizzo di quel canale della morte. Per i migranti economici, invece, è giusto e doveroso sensibilizzare i Paesi d'origine al fine di evitare che finiscano vittime della tratta di esseri umani e che si trovino a rischiare la vita per finire spesso in situazioni di instabilità sociale ed economica: esistono i canali legali che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro proprio per scongiurare la precarietà. Inoltre, il provvedimento fornisce ulteriori strumenti per contenere la pressione migratoria, anche in un'ottica di tutela delle frontiere esterne e di prevenzione di potenziali rischi di infiltrazioni da parte di soggetti contigui alle organizzazioni terroristiche, alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. Concludo dunque, signor Presidente, nel dire che, per questi motivi, riteniamo necessario che il provvedimento sia attuato in tempi brevi per proseguire su una linea politica che riporti al centro il rispetto

del Governo, colleghe e colleghi, è un momento particolare quello di oggi in quest'Aula, perché andiamo ad approvare un provvedimento che credo andrà nella direzione giusta. Si è tenuta una ampia discussione in Commissione e voglio ringraziare il presidente Vito Petrocelli, sia per il garbo che per

nei confronti della Libia, con la cessione a titolo gratuito di dodici importanti imbarcazioni, ma è anche un atto nell'interesse dell'Italia stessa, e direi dell'Europa, perché ci poniamo finalmente in contrasto rispetto all'immigrazione clandestina, in sintonia con quello che è stato anche il programma del centrodestra. Ho piacere che quest'oggi in Aula

di evidenziare l'importanza di contrastare queste partenze. Tutti coloro che mi hanno preceduto lo hanno evidenziato, anche con enfasi e con forza, e seguendo, mi permetto di dire, un elemento reale: abbiamo avuto migliaia e migliaia di morti nel Mediterraneo. È successo tutto per caso? Soprattutto, davanti alle coste libiche sembra quasi che ci troviamo di fronte al triangolo delle Bermude. Era un caso? Come mai sono avvenuti questi affondamenti di imbarcazioni, che non sono assolutamente adatte per il trasporto di esseri umani (peraltro, provenienti dalla Cina per una rotta che perfettamente conosciamo)? Abbiamo citato l'operazione Sophia. L'ammiraglio Credendino nella precedente legislatura, sentito nelle Commissioni esteri e difesa, ebbe a dire che in questo tipo di operazione vi è anche la possibilità di controllare i natanti e di fare dei controlli su quelle imbarcazioni. Allora, visto che abbiamo la possibilità di avere il Governo presente, credo che sarebbe opportuno incominciare a pattugliare con le imbarcazioni nostre nazionali, ma anche con quelle estere che fanno parte di questa operazione, e avviare un contrasto per verificare come mai questi gommoni, tutti grigi, che vediamo nelle immagini televisive, arrivano nei porti

dovremmo probabilmente prevedere l'impiego, con l'intervento anche dell'Italia, di imbarcazioni diverse. Mi riferisco, ad esempio, a gommoni da diporto di 13, 14 o 15 metri, dotati di due motori, che possano consentire di pattugliare le coste libiche, perché non dobbiamo mai dimenticare che ci troviamo di fronte a 1.770 chilometri di costa, non semplici da pattugliare. Con queste imbarcazioni, allora, possiamo fare tanto. Mi auguro che anche i tempi di preparazione degli equipaggi siano celeri. Mi rendo conto della difficoltà, soprattutto e in particolare per l'utilizzo delle due imbarcazioni provenienti dalla Guardia di finanza. Mi riferisco a quelle da 27 metri, che sono dotate, non solamente di sofisticati sistemi *radar* che possono essere utilissimi, ma che hanno anche una avanzata tecnologia, soprattutto nella carena. Un collega, Un collega, prima, ricordava la possibilità di arrivare fino a 43 miglia, che è una velocità considerevole per un'imbarcazione di quella portata, che ha una velocità di crociera di 21 nodi, ma riesce a mantenere anche le 43 miglia. Possiamo quindi efficacemente intervenire

su 100 che arrivano, più di 90 non avrebbero alcun titolo e alcuna ragione per rimanere in Italia. Se vogliamo allora aiutare veramente chi ha il diritto - e noi abbiamo il dovere di accogliere chi si trova in determinate situazioni gravissime: le mamme, i bambini, coloro che davvero fuggono dalla guerra - dobbiamo incominciare a porre un contrasto forte nei confronti di coloro che vengono qui molto spesso semplicemente per saccheggiare lo Stato sociale. Questa è la verità. Vogliamo farlo - e credo che possiamo - tutti insieme, anche in quest'Aula con questo inizio di operazione molto importante, che non si potrà certamente fermare qui. Il nostro vice presidente Tajani, nel corso di un recente incontro, ha parlato di un grande piano per l'Africa, al quale dovrebbero contribuire tutte le Nazioni che hanno la possibilità di farlo; cercare di aiutare quei Paesi a incominciare a lavorare, in particolare, nell'agricoltura.

con unità di controllo *radar* e soprattutto con droni che riescano a intercettare le imbarcazioni che partono. Questo dobbiamo incominciare a fare. Esprimiamo un voto naturalmente favorevole, anche in ossequio ai principi che abbiamo seguito, quelli del Trattato di Bengasi del 2008, poi entrato in vigore nel 2009 e che portava le firme di Gheddafi e del *premier* di allora Silvio Berlusconi, che aveva preconizzato ciò che sarebbe accaduto. Da quel momento

il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire è stato accolto positivamente, come abbiamo visto, da tutte le forze politiche sia di maggioranza che di opposizione. D'altra parte, esso si inserisce nell'alveo di una continuità con quanto è stato fatto anche nelle precedenti legislature. È un provvedimento che fornisce un aiuto importante alle diverse strutture libiche - sembra siano almeno tre - che, a vario titolo, sono competenti e responsabili in tema di polizia e soccorso marittimo. In termini generali, però, occorre prendere atto della situazione, secondo me, e riflettere su un punto: bisogna chiedersi se sia opportuno continuare a interloquire con il solo al-Sarraj, o se sia meglio allargare l'interlocuzione ad altri attori. Non è inutile, infatti, ricordare che già nel luglio dello scorso anno il presidente francese Macron aveva invitato a Parigi sia al-Sarraj sia Haftar. Successivamente, nel maggio di quest'anno, la Francia ha convocato una nuova conferenza che ha visto la partecipazione, oltre che di al-Sarraj e di Haftar, anche del presidente della Camera dei rappresentanti La Francia quindi evidenzia una strategia di ampio respiro rispetto a quella un po' più angusta adottata dall'Italia degli anni recenti, laddove ci si era concentrati soltanto sulla figura - decisiva, sicuramente - di al-Sarraj, trascurando gli altri soggetti che invece potrebbero avere un ruolo importante anche nel contrastare i traffici traffici di coloro che sfruttano la tragedia dei migranti e dei naufragi. Con il decreto-legge in discussione - è stato ricordato - si cedono dieci unità navali costiere da 11 metri e due unità navali da 27 metri. da 27 metri. Le dieci piccole unità sono unità di polizia marittima che la Guardia costiera e la Capitaneria di porto utilizzano per la vigilanza e queste possono navigare con mare calmo o mare appena formato, mentre i due pattugliatori d'altura della Finanza sono unità che hanno grande autonomia. È altresì previsto un periodo adeguato e congruo di familiarizzazione degli equipaggi libici per la conduzione di queste motovedette. Le piccole sono sostanzialmente dei motoscafi, quindi non c'è bisogno di una lunga fase di familiarizzazione: ventotto giorni sono più che sufficienti.

Per queste unità era già prevista la sostituzione. Attualmente, tra l'altro, non sono - tranne forse qualche caso sporadico - impiegate in compiti operativi.

anche di altri fattori, a mio parere. In primo luogo, abbiamo visto che i migranti vivono nel terrore e nella disperazione dell'eventualità di essere riportati indietro, laddove, come hanno

che molti di loro hanno subito torture e violenze feroci, anche perché la Libia affida la gestione dei soccorsi alle stesse autorità che poi portano i migranti nei famigerati centri di detenzione e quel Paese non offre, com'è stato detto, garanzie per l'incolumità dei migranti intercettati o dei naufraghi salvati in mare, né consente accoglienza e accesso a una procedura d'asilo. Inoltre, sebbene risulti formalmente istituita una zona SAR libica, come veniva ricordato dalla collega, affinché il servizio di soccorso sia effettivo è necessario che lo Stato sia in grado di garantire continua operatività, coordinata ed efficace, dei servizi SAR, che istituisca un centro e sottocentri di soccorso e di coordinamento e che disponga di personale adeguato quantitativamente e qualitativamente (cosa che si sta facendo ma non è ancora completata). Tutto il servizio deve essere integrato in uno specifico contesto normativo, quindi la cessione delle motovedette ai libici è un primo passo cui si deve aggiungere una serie di iniziative e misure volte a creare un flusso - come veniva anche raccomandato - regolato e sicuro di migranti verso l'Europa, al quale si dovranno affiancare corridoi umanitari per i richiedenti asilo. Sotto un altro aspetto, occorre tener presente il dato economico. Va rilevato, cioè, che attualmente le rimesse dei migranti verso i Paesi d'origine superano di gran lunga i contributi allo sviluppo stanziati dall'Europa.

Abbiamo tutti negli occhi lo sguardo terrorizzato di Josefa e dobbiamo capire che quel terrore supera anche la paura di morire in mare. Chi parte è consapevole di mettere a rischio la propria vita, ma è certo che, da dove parte, non esiste possibilità di vita. Concludendo, siamo di fronte ad un decreto-legge che ha molti aspetti positivi e che va rapidamente convertito in legge. Tuttavia, non basta ancora.

proprio questa continuità, in un contesto sempre più pesante e sempre più esasperato, che a mio avviso va interrotta e va ripensata. Va interrotta, perché se andiamo un po' sotto il linguaggio diplomatico, non stiamo affatto collaborando con il Governo al-Sarraj, che non esiste: non si può collaborare con un'entità che non esiste. Sapete perfettamente, come me, che il Governo al-Sarraj non controlla neanche il palazzo in cui sta; sapete perfettamente che la Libia è fatta di due Stati, tre Parlamenti e di centinaia di milizie, che sono le uniche che, in lotta le une con le altre, controllano il territorio. Quindi, di fatto, noi stiamo - anzi, voi state - continuando a rafforzare le milizie, che si spartiranno queste motovedette, che non servono per salvare nessuno: sono motovedette di circa 10 metri e non si fa salvataggio in mare in questo modo, come è evidente e come ricordava il collega. Dunque state semplicemente rafforzando le milizie libiche, che si spartiranno queste motovedette, come già si spartiscono il commercio in nero del petrolio (che pare non interessi a nessuno) il commercio della droga (che effettivamente interessa ancora meno) e altri traffici illeciti, che non sono gestiti né da Haftar, né da al-Sarraj, ma dalle milizie libiche, con alleanze molto volatili e molto fragili.

di partenza da Sabratha a Garabulli e a Zuwara. Pensate davvero di prosciugare un oceano con un secchio?

sono una che pensa che la regola, la legge e le convenzioni internazionali siano l'unico modo di convivenza civile. terzo elemento: le convenzioni internazionali non parlano di porti sicuri, ma di posti sicuri

persino la Commissione europea e le testimonianze univoche di centinaia, di migliaia di profughi, che hanno un unico racconto da fare: stupri, violenze e torture. Le avete viste come me, ne avete visto i *reportage,* le foto, eccetera. Anche se avete cuore di rimandare la gente che scappa in questi posti, io non credo che sia una grande prospettiva, una grande politica e neanche una grande visione.

di certo il nostro «lontano dagli occhi, lontano dal cuore» con l'espulsione anche delle navi delle organizzazioni non governative aiuta questa schizofrenia totale. Infine, se oltre alla sofferenza e al dolore di queste persone che hanno l'unico demerito di avere una pelle di colore diverso dalla nostra,

ci risparmiassimo gli insulti ci faremmo un favore. Voi sapete come me che non c'è pacchia che tenga; voi sapete come me che non sono in crociera; voi sapete come me che non ci sono i taxi del mare voi sapete come me e come i nostri nonni che sfuggono dalla miseria e dalla fame, in cerca di una possibilità di vita migliore.

così, non è neanche aperto. Gli altri non sono neanche visitabili: nove o dieci sono visitabili dall'UNHCR, ma le centinaia di altri luoghi privati di tortura, di stupro, di violenza non sono visitabili da nessuno. Non credo sia una grande politica. Penso invece che l'apertura di canali legali, l'apertura di scambi richiesta di approvazione delle convenzioni internazionali sarebbe più utile, più efficace.

Non si svuota un oceano con un secchio. La mobilità è globale e non la fermerete certamente voi.

ma contavo sulla vostra personale cortesia democratica. Non è possibile che un'unica o pochissime pochissime voci che sono in disaccordo debbano ottenere minacce, insulti e mancanza di rispetto anche in quest'Aula. Ho concluso, signor Presidente, ma vi ricordo che non siete nella curva Sud, ma nell'Aula più alta delle istituzioni democratiche di questo Paese! Voi dovete dare l'esempio di compostezza istituzionale, di rispetto per le opinioni diverse. *(Proteste dei Trattenete gli insulti. Ha detto qualcuno molto più importante di me che gli insulti qualificano chi li fa, non chi li riceve.

Fratelli d'Italia è assolutamente d'accordo con questo provvedimento che in piccola parte rafforza anche la Guardia costiera libica, di conseguenza limita in parte la partenza dei barconi e quello che ne consegue. Stiamo faticosamente cercando di rimediare ai danni che ci sono stati in questi anni. Negli ultimi sette anni i rapporti tra noi e la Libia sono completamente cambiati: siamo passati dall'Accordo di amicizia e cooperazione di Bengasi del 2008, quando l'Italia e la Libia dialogavano sotto tutti gli aspetti, controllavano i confini e non c'erano sbarchi in Italia, a una situazione nel 2011 di guerra alla Libia, guerra a Gheddafi e caos totale in Libia, dal quale è derivato

solo il 15 per cento con le caratteristiche per avere la qualifica di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra e poco

scappavano da condizione di vita proibitive, questo sicuramente, ma non erano rifugiati. Come siamo arrivati a questo? Ci siamo arrivati - le responsabilità prima o poi dovranno essere chiarite - con un attacco alla Libia voluto dalla Francia per togliere all'Italia il rapporto privilegiato che aveva e accordi energetici molto interessanti (era questo che preoccupava particolarmente la Francia). Il fatto che la Francia abbia compiuto un atto ostile a carattere militare nei confronti dell'Italia è un fatto gravissimo, ma è ancora più grave che qualcuno in quei giorni abbia sostenuto l'intervento francese dentro le nostre istituzioni fino ai livelli più alti. Si tratta di una responsabilità di tradimento degli interessi nazionali di cui la storia prima o poi

Fratelli d'Italia lo ha sempre detto in modo molto chiaro: l'unica soluzione è un blocco navale al largo delle coste libiche in accordo con le autorità libiche; su questo mi unisco a delle considerazioni che sono state fatte dai miei colleghi prima di me. La Libia non è controllata dal Governo al-Sarraj e non è governata dal Governo di Tripoli. Ripeto, occorre un blocco navale in accordo con le autorità libiche e con chi controlla le coste dalle quali partono i barconi; un blocco navale che impedisca la partenza dei barconi, le morti in mare e l'enorme ingiustizia di una immigrazione incontrollata. Qualcuno prima di me ha parlato di attivare canali legali di immigrazione: è giustissimo. L'immigrazione deve essere gestita con dei canali legali. D'altronde, in Italia esiste il sistema del decreto flussi, che ogni anno stabilisce quante persone possono entrare e da quali Paesi. I decreti flussi sono stati azzerati negli ultimi anni e ciò è una vergogna perché tutta la quota di immigrazione è stata colmata con l'immigrazione illegale. Questo è inaccettabile, perché non si capisce in nome di cosa un peruviano che voleva venire in Italia non poteva farlo perché i decreti flussi non lo permettevano, mentre qualcuno che pagava gli scafisti poteva arrivare illegalmente in Italia. Si arriva poi alle situazioni grottesche

per i venezuelani. Avrete sentito tutti la situazione drammatica del Venezuela. I venezuelani scappano nelle Nazioni vicine, prima fra tutte la Colombia. Perché un venezuelano non deve avere il diritto di canali diretti?

La prima riguarda il costo di questa operazione. Il decreto-legge parla di un costo complessivo di 2.520.000 euro, però non è esatto. Abbiamo chiesto al Governo, che ce li ha forniti, i dati del valore inventariale dei mezzi. Il valore inventariale dei mezzi ammonta, in totale, a 642.000 euro. Quindi, il valore dell'operazione è pari a circa 3.100.000

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ritorno sul provvedimento che oggi stiamo discutendo. Si tratta di un provvedimento che persegue una strategia di continuità con quanto fatto dai Governi precedentemente in carica, ossia cercare di aiutare l'instaurazione di una statualità della Libia che che vediamo, purtroppo, essere molto latente e che fa emergere situazioni di criticità enormi, come contrasto alla criminalità organizzata ed internazionale e per prevenire potenziali rischi di infiltrazione di soggetti contigui alle organizzazioni terroristiche.

traversata del deserto sahariano. Richiamo tuttavia l'attenzione del Governo sul fatto che con questo decreto-legge viene affrontato solo il problema finale del più complesso fenomeno migratorio in atto nel Mediterraneo centrale, ovvero, il rafforzamento della Guardia costiera libica, che - come purtroppo si è capito dagli ultimi avvenimenti -

che ringrazio veramente di cuore - in un'intervista ha ribadito che su questo punto la normativa è chiarissima: «Noi continuiamo ad operare secondo quelle che sono le convenzioni internazionali del mare». In sostanza, chi riceve la chiamata, «deve operarsi subito affinché quella persona o quella nave in pericolo possano

senza dire con quali fondi avrebbe sostituito queste motovedette. Quindi la notizia del decreto-legge pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 10 luglio ovviamente ha destato molta preoccupazione nelle diverse marinerie, tra le quali ribadisco ci sono anche quelle di Goro e Gorino che rimangono sguarnite. Come ha

Cari colleghi, non è semplicissimo intervenire in questo dibattito perché naturalmente, come sempre capita quando si parla di temi così delicati e quando si parla di Libia, un conto è il voto che noi siamo chiamati a dare, un conto è l'analisi che siamo chiamati a fare, un conto sono le sensibilità diverse che attraversano il nostro Parlamento.

e perché è giusto dotare di un equipaggiamento navale le forze di controllo costiero libico.

Purtroppo lo sapevamo un po' tutti in quest'Aula che non esiste la statualità libica. Sappiamo addirittura che c'è un Governo, quello di Haftar, che con la collaborazione di statualità estere e anche europee ha lavorato in questi anni per arrivare ad una tripartizione della Libia, nonostante la comunità internazionale abbia insediato un Governo che noi sempre abbiamo appoggiato, con Letta, con Renzi, con Gentiloni Silveri oggi con il Governo Conte in uno spirito di continuità, perché era il Governo legittimato dall'ONU. Ma questo Governo controlla la Libia? Scusate, non siamo su «scherzi a parte», lo sappiamo benissimo che questo Governo non controlla la Libia. Sappiamo benissimo che non la controllano neanche gli altri due Governi. Sappiamo benissimo che ci sono dei soggetti tribali municipali che non a caso sono stati al centro del lavoro che nei mesi scorsi ha fatto il Governo

Un conto allora è il mondo che vorremmo vivere, un conto è il mondo che viviamo perché la politica estera non è un pranzo di gala e noi, purtroppo, dobbiamo fare i conti con quello che c'è non con quello che vorremmo che ci fosse. Ho sentito prima alcuni colleghi che hanno detto che chi arriva non ha i documenti. ma volete che vadano a chiedere il certificato penale a Mogadiscio quando partono da realtà che sono devastate, prive di qualsiasi statualità? Allo stesso modo, non ci meravigliamo, purtroppo, di quello che la senatrice Bonino ha dichiarato che, se mi consentite, non può essere un elemento di divisione di questo Parlamento: sappiamo tutti che i diritti umani, per come noi li concepiamo, non sono adeguatamente rispettati in Libia. Sappiamo benissimo che nei campi di detenzione - a volte non sappiamo nemmeno chi detiene chi

dovrebbe fare, però, il Governo di un Paese come l'Italia? Che cosa dovevano fare i Governi precedenti? Non dimentichiamo, infatti, e lo ha detto anche il ministro Salvini (avrei avuto piacere che lo dicesse di più ma comunque l'ho sentito, per cui l'ha detto),

È bello o brutto ridurre gli sbarchi? Colleghi, cosa volete che vi diciamo? È l'unica strada possibile oggi perché noi rischiamo, se non seguiamo la via di dare più ordine agli arrivi nel nostro Paese, di veder nascere razzismo tra le classi popolari di questo Paese che si vedono insidiate dall'arrivo sconclusionato e scomposto dei migranti. Non è un problema di destra o di sinistra, è un problema di buon senso. Tutti noi sappiamo di essere orgogliosi di ciò che fa la Guardia costiera italiana, di quello che fanno i militari italiani, dei salvataggi che, dal Governo Letta in poi, in linea di continuità tutte le forze militari italiane hanno fatto; e vogliamo che continuino a fare. Siamo rassicurati da ciò che ha detto il ministro Moavero Milanesi ieri: vogliamo che si continuino a salvare vite umane ma, nello stesso tempo, non possiamo non porci il problema di cercare di regolare questo fenomeno. Se non lo regoliamo, infatti, ne saremo inevitabilmente sommersi e - aggiungo io ne saranno sommerse le forme democratiche come noi le concepiamo nelle società occidentali ed europee. Dunque, lasciamo perdere queste dieci motovedette: è ovvio che noi non possiamo che dare un parere positivo.

che arriva dal Mar Mediterraneo in modo travolgente anche per le questioni demografiche. Sappiamo tutti, infatti, di aver bisogno degli extracomunitari, ma sappiamo anche di avere qui, tra i banchi del Parlamento, persone che vengono da Paesi diversi e che si sono integrate secondo un ordine e un rispetto delle regole che è esattamente quello che noi vogliamo per tutti coloro che arrivano qui come punto di unione nazionale. ero Presidente della Camera, eletto dal centrodestra, e mi dichiarai favorevole, quindici anni fa, allo *ius soli*. Nessuno disse niente, perché allora lo *ius soli* non era elemento divisivo come è diventato quindici anni dopo. Siamo andati avanti o siamo andati indietro? Siamo andati indietro, purtroppo.

La politica si fa col cuore e con la mente. Noi dobbiamo farla col cuore, col cuore salviamo le vite umane e con il cuore cerchiamo di dare solidarietà. Io ricordo quando andai a Lampedusa la polizia mi chiese se volevo entrare in una casetta. Entrai in una casetta dove c'erano tre somali: papà, mamma e una bambina. avevano perso tre figli nella traversata. Erano partiti da Mogadiscio con quattro figli ed erano rimasti con una bambina che, sperduta, aveva un giochino con cui si trastullava. Questi due genitori avevano gli occhi che guardavano nel vuoto. Ebbene queste tragedie sono la catena di tante tragedie che, dalla Turchia alla Grecia a Lampedusa ad altre parti dell'Europa, noi possiamo vivere tutti i giorni. Noi dobbiamo essere intrisi di senso di umanità ma, avendo

anche per fare in buona fede delle cose buone, di produrre dei pessimi risultati. Dunque, il voto a favore e di condivisione su questo decreto-legge va oltre, per il Gruppo Per le Autonomie, il

e anche ai problemi di questa nostra Italia, che vuole coniugare umanità e legalità.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, sono onorato di intervenire per la prima volta in questa Aula ed in particolar modo di farlo oggi in merito ad un provvedimento riguardante la sicurezza delle nostre coste. Va detto subito che il provvedimento in esame persegue l'idea di affidare alla Guardia costiera libica il controllo delle proprie coste e, a tal fine, prevede qualcosa di concreto per ottenere tale scopo. I libici hanno interesse ad avere il controllo delle proprie coste e delle proprie acque territoriali. L'Italia ha attenzione a che, in conseguenza di un più puntuale controllo delle coste libiche, partano meno imbarcazioni. Meno partenze significa soprattutto - che è la cosa che ci sta più a cuore - meno persone a rischio di morire. Come abbiamo visto, infatti, alcune imbarcazioni fatiscenti, ovvero preda delle condizioni del mare inclemente, ma anche, ove trattasi di scafi affidabili, con un carico smisurato di persone, finiscono ben presto in modo tragico la propria traversata. Il Mar Mediterraneo ha inghiottito 30.000 persone negli ultimi quindici anni: un'intera città deglutita da un mare incolpevole. Le speranze di una vita migliore sono finite per questi uomini, donne, ragazzi e bambini, prima ancora di mettere piede sulla terra tanto agognata. Molti scappano dai propri Paesi a causa delle guerre o di terribili condizioni che azzerano i loro diritti civili o le loro libertà. tuttavia, che partano mettendosi nelle mani di mercanti di uomini a cui non interessa nulla del loro destino. Le partenze vanno fermate, ma non vanno fermati gli arrivi. Chi ha diritto a ottenere una protezione internazionale, che è disciplinata dal diritto internazionale e dal diritto europeo, deve poter raggiungere l'Europa - lo ripeto, l'Europa - in modo sicuro. I corridoi umanitari devono essere aperti per i rifugiati. Chi ha diritto a un permesso di soggiorno in quanto rifugiato deve poter raggiungere il territorio europeo in modo dignitoso e deve essere accolto come un fratello. Quello di cui non abbiamo assolutamente bisogno è una migrazione irregolare che non distingua tra chi ha diritto e chi non può accampare alcun diritto. II rispetto del diritto è alla base di ogni civiltà; se mancasse questo, verrebbe meno il nostro stesso stato di diritto. Purtroppo la migrazione irregolare, oltre a causare le 30.000 vittime stimate, che potrebbero addirittura essere di più, ha innescato nel nostro Paese un aumento della percezione dell'illegalità. Alla base dell'accoglienza ci deve essere anche il lavoro per tutti e l'idea che le persone che accogliamo possano costituire nuclei familiari nel nostro Paese. Questo modello è lo stesso che ha visto protagonisti i nostri bisnonni emigranti a inizio secolo, poi i nostri nonni e in alcuni casi i nostri padri - perché anche negli anni Sessanta ancora si emigrava - e che oggi vede protagonisti anche i nostri figli. Avvalorare l'idea che l'Italia possa, o addirittura debba, accogliere tutti è una follia; diventa una politica improponibile soprattutto per due ordini di motivi. Il primo è che ormai tutti sappiamo che le partenze sono gestite da autentici delinquenti, da mercanti di uomini dei giorni nostri. Il secondo è che non possiamo permetterci di ospitare quasi 200.000 persone ogni anno, posto che quattro su cinque tra i migranti accolti non hanno diritto a essere ospitati secondo le regole europee. Non possiamo fare finta che, una volta negato il permesso di soggiorno, i migranti non si diano alla clandestinità. Si stimano più di 600.000 clandestini, con ovvie implicazioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. Non possiamo nemmeno fare finta che l'Italia possa sostenere da sola l'integrazione di tutti coloro che ne hanno diritto. In termini di bilancio pubblico, non possiamo distogliere quasi 5 miliardi annui per la gestione dei migranti, quando dobbiamo fare i conti coi saldi di bilancio e abbiamo innescato politiche di austerità nei confronti dei nostri cittadini. Ecco perché la politica deve innanzi tutto porsi il problema di fermare le partenze dalla Libia, per smaltire nel migliore dei modi le pratiche relative ai migranti già presenti. Il decreto-legge al nostro esame è certamente rispettoso delle prerogative del Parlamento. Non è il primo provvedimento in tema, ma va relazionato alle politiche di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia, già intraprese dal Governo Berlusconi nel 2009 per arginare i flussi migratori e tutelare gli interessi italiani in Libia. Sto rammentando il cosiddetto Trattato di Bengasi, cioè il Trattato di amicizia e cooperazione tra Italia e Libia, sottoscritto dal presidente Berlusconi e da Gheddafi il 30 agosto 2008, che fu ratificato dall'Italia il 6 febbraio 2009. Con il Trattato di Bengasi si raggiunse un risultato storico tra i due Paesi e si chiuse un contenzioso che si trascinava dagli anni del Dopoguerra. Va ricordato che, dopo quell'accordo del 2008, in Libia cessò la celebrazione del giorno della vendetta, indetto da Gheddafi il 7 ottobre del 1970 in ricordo della ritorsione anti-italiana. Sul tema del contenzioso Italia-Libia, Forza Italia ha presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo in Commissione esteri, con il quale impegna l'Esecutivo ad affrontare l'irrisolta questione dei crediti storici vantati da oltre vent'anni da oltre 100 imprese italiane nei confronti di enti e amministrazioni libiche, per un importo complessivo di più di 200 milioni di euro. Questi crediti erano stati riconosciuti dal Governo libico nel 2013 e 2014 sulla base del negoziato avviato nell'ambito del Comitato crediti, come previsto dal Trattato di amicizia. Ma, per tornare al tema del decreto-legge, non è la prima cessione di motovedette alla Guardia costiera libica. Così come i nostri ufficiali e sottufficiali si sono già adoperati per addestrare e formare gli addetti libici. Nel 2009 furono cedute tre motovedette, tre nel 2010, altre le abbiamo riparate. Due motovedette sono state affondate nel 2011, durante l'attacco francese (noto come attacco della coalizione occidentale). Poi, più di recente, nell'aprile 2017, il ministro Minniti aveva consegnato altre quattro motovedette, investendo nella formazione della Guardia costiera e della Marina libica. Quindi la cessione di dodici unità navali prevista dal provvedimento in esame, a titolo gratuito, va nel senso auspicato di un più puntuale intervento libico nella propria area SAR. Sono assicurate, altresì, le risorse finanziarie necessarie per garantire la manutenzione e l'addestramento del personale. Del resto, si tratta di somme irrisorie rispetto agli enormi oneri affrontati in questi anni per gestire il complesso fenomeno migratorio. Lo scopo è quello di incrementare la capacità operativa della Guardia costiera e della Marina libiche per contrastare i traffici di esseri umani e per le attività di soccorso in mare. Le controversie sul ruolo delle ONG non possono che diminuire se aumenta il controllo delle aree di soccorso e salvataggio in mare da parte dei libici. Le frontiere italiane del Mediterraneo sono quelle europee, di questo deve farsi persuasa la Commissione europea. Ma se l'Italia, se noi dimostriamo concretezza e serietà nel gestire il fenomeno migratorio illegale e al tempo stesso la volontà a non fermare l'accoglienza di chi ne ha diritto, anche l'Europa dovrà farsene carico.

*(M5S)*. Signor Presidente, colleghi e colleghe, Governo, le donazioni di imbarcazioni per il pattugliamento e il salvataggio in mare alla Guardia costiera e alla Marina libiche sembrano giocare specularmente la battaglia politica italiana. Circa venti giorni fa, il portavoce della Guardia costiera libica asseriva a un'agenzia giornalistica italiana, forse suggestionato da qualche politico oggi all'opposizione, che il nostro Governo non sarebbe stato in grado di offrire alle autorità libiche alcuna imbarcazione idonea ad affrontare i natanti degli scafisti. Anzi, con sarcasmo affermava che al massimo il nostro Governo avrebbe fornito alla Guardia costiera nordafricana solo qualche gommone. Probabilmente, la fonte del portavoce della Guardia costiera libica sperava in un rifiuto aprioristico delle autorità libiche. Oggi leggiamo, invece, che le imbarcazioni offerte sono di tutto riguardo e ve ne sono un paio che superano abbondantemente i 20 metri. Cosa significa ciò? Significa che, dopo aver addestrato le forze libiche, le stesse potranno controllare le loro loro acque territoriali, avranno la forza di interdizione nei confronti di scafisti e contrabbandieri in generale, iniziando così a considerarsi uno Stato sovrano. È chiaro che, in questo ordine regionale, alcuni Paesi cerchino di non emancipare le Forze armate libiche, così come risulta limpido il gioco di alcune opposizioni parlamentari italiane che, trascurando gli affari italiani e dei migranti e facendo sponda con pezzi dell'Esercito e dei guardacoste libici, cerchino di impedire qualsivoglia cambiamento in quello scacchiere. Per quanto riguarda le spese, si può tranquillamente affermare che la missione dei militari italiani costi meno della missione delle Forze dell'ordine in un qualsiasi centro di identificazione ed espulsione (CIE) un centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), siti in territorio italiano. Per esempio il CARA di Mineo, in provincia di Catania, impiega ogni giorno giorno 100 poliziotti, che provengono da tutte le questure d'Italia e dai vari reparti mobili sparsi sul territorio. Ad ognuno di questi operatori viene garantito alloggio e pasto in *hotel*, più lo straordinario giornaliero e il trattamento di missione. Mediamente per un singolo poliziotto si spendono 200 euro al giorno oltre lo stipendio. Se si moltiplica questo importo per il numero dei poliziotti impegnati, la spesa risulta di 20.000 euro al giorno, che moltiplicati per 365 giorni. Vi rendete conto? Basterebbe chiudere uno degli innumerevoli CIE o CARA italiani per pagare l'intera PD)*. In sostanza, per garantire la sicurezza al CARA di Mineo si spendono complessivamente circa 9 milioni di euro l'anno. Se l'invio di queste motovedette riesce a ridurre gli sbarchi e a portare alla chiusura di un solo centro in Italia, il Governo italiano può tranquillamente affermare che questa operazione è a costo zero. Inoltre Inoltre è bene ricordare che qualche giorno fa il Consiglio europeo ha accettato la proposta del Governo libico di estendere la zona di *search and rescue* (SAR) per le autorità marittime della Libia. Ormai si va oltre le fatidiche 12 miglia. Quindi, se da una parte concordiamo con i libici il controllo di uno specchio di mare, che va ben oltre le acque nazionali, dall'altro non possiamo esimerci dal fornire loro le motovedette d'altura. In ogni caso, la fornitura prospettata è un primo significativo passo in questa direzione. Un passo al quale, spero, ne seguano altri, magari con la fornitura di ulteriori motovedette classe 300, più consone per il salvataggio in mare, oltre che provviste di sistema di raddrizzamento. Inoltre, vi vorrei segnalare che nel SAR, come definito precedentemente, lo Stato di Malta, si sia fatto accordare un tratto di mare corrispondente a 650 volte l'estensione dell'isola, quasi sempre ha delegato altri ad effettuare i salvataggi e quasi mai ha accettato l'arrivo dei naufraghi nei propri porti.

sia squisitamente politico, per portare quel Governo a firmare tutti gli accordi per la tutela dei diritti umani, primi fra tutti quelli dei migranti. Abbiamo degli obblighi verso quel Paese: dobbiamo aiutarlo a rientrare fra i Paesi stabilizzati. Per quanto riguarda gli accordi tra l'Italia e la Libia, è bene ricordare che la prima bozza di Trattato fu sottoscritta dal Governo Prodi, il comunicato congiunto, nel 1998, con Gheddafi, proprio per impegnare il colonnello a contrastare il nascituro terrorismo integralista e, soprattutto, per favorire le estrazioni Nel 2008, con il Trattato di Bengasi, il Governo Berlusconi chiuse l'accordo sostanzialmente in tre punti: oltre al punto già citato, si impegnava il Governo libico a contrastare il il fenomeno dell'immigrazione, che già mostrava la fisionomia di un vero e proprio esodo. Torniamo però al primo punto dell'accordo del 2008, in cui si impone ai contraenti di non ricorrere ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica della parte opposta. Cosa che noi, anzi voi che che stavate seduti tra questi banchi avete disatteso nel 2011, prima votando a favore dell'uso delle basi NATO per bombardare la Libia, poi entrando direttamente nel conflitto. *(Commenti dal Gruppo

quali furono i partiti che votarono a favore della guerra in Libia. Votarono a favore il PdL, partiti minori e il PD; votarono contro la guerra la Lega e l'Italia dei Valori. Dico questo per ribadire che lo spirito di collaborazione del nostro Governo con il riconosciuto Governo libico non intende proseguire, come alcuni colleghi affermano, la vecchia politica bilaterale con la Libia. Di quella politica dovremmo solo vergognarci. Solo Solo affermare che ci sia continuità tra noi e voi vi conferirebbe uno *status* che voi non meritate. *(Applausi

Signor Presidente, io intendo replicare per un motivo molto semplice. Io stesso ammetto di essermi abbastanza annoiato durante la mia relazione introduttiva sul provvedimento, ma fortunatamente il dibattito poi si è sviluppato su toni politici che apprezzo molto. Vorrei iniziare, per replicare ad alcune delle posizioni espresse in maniera squisitamente politica in quest'Aula, da uno degli ultimi interventi, quello del senatore Casini. Senatore Casini, Casini, ascoltare la sua citazione di Mao Tse-tung, quando ha detto che la politica estera non è un pranzo di gala, non ha davvero prezzo, ma per il resto il suo intervento

per una questione che tutti quanti noi conoscevamo e conosciamo. Mi riferisco cioè al fatto che la Libia è divisa in tre unità statuali, che ci sono parti della Libia controllate da milizie, come ricordava anche la senatrice Bonino, che non è

se ce le portiamo dietro da molti anni, quantomeno dal 2011, quando i nostri alleati, soprattutto la Francia ma anche altri alleati NATO, probabilmente non si sono comportati proprio come se fossero nostri alleati

la senatrice Bonino ha sollevato delle questioni rilevanti. Mi dispiace soprattutto che abbia paragonato questo intervento all'attività di un secchio che non può svuotare l'oceano. A me sembra ingeneroso nei confronti del provvedimento in esame che - lo ripeto - non ha alcuna ambizione di controllare situazioni molto più grandi, ma è come la marea e se non la contrasti non la puoi fermare. È come se potessimo dire che con l'innalzamento di un grado della temperatura globale non si alzasse il livello del mare e non si debba intervenire. Anche l'intervento di un secchio ha un suo effetto sull'Oceano e soprattutto sul Mediterraneo, mi permetto di dirlo. Vorrei altresì ricordare al collega De Falco, che pure ha sottolineato in maniera giusta, che si danno motovedette e si formano persone per intervenire in una parte della Libia dimenticandosi dell'altra parte: la parte controllata da Haftar,

non partono barconi dalla parte controllata da Haftar. Se partono dalle coste libiche controllate dal Governo di Tripoli, è a quest'ultimo che dobbiamo fornire anche un solo secchio per controllare quelle partenze. faccio un richiamo alla corretta interpretazione fatta da senatori e senatrici sull'utilizzo di queste imbarcazioni, che vengono sottratte ad alcune Capitanerie di porto. Già in Commissione il sottosegretario Molteni si è espresso su questo argomento, ma io voglio sottolineare un piccolo particolare: da sinistra, con la senatrice Boldrini, fino a destra, con un senatore di Forza Italia, è stato detto che

lo diceva la senatrice Boldrini. Però questo messaggio e questo *slogan*, ossia pensiamo prima alle vongole di Goro e Gorino, cioè pensiamo prima agli italiani, non mi pare che sia proprio uno *slogan* del Partito Democratico;

dare anche solo con un secchio la possibilità di fermare ondate migratorie e il traffico di esseri umani significa pensare prima di tutto agli italiani.

solo per ricordare che con l'emendamento 1.1 noi ci limitiamo ad inserire nel decreto-legge, peraltro in prima lettura, quello che il Governo assicura in modo verbale. Non comprendiamo perché il Governo non debba assicurarlo nel decreto-legge attraverso l'accoglimento del nostro emendamento che si limita a dire che devono essere salvaguardati i livelli di efficienza e di capacità operativa delle Capitanerie di porto, Guardia costiera e Guardia di finanza interessate. Se il Governo è d'accordo con questo principio, inseriamolo nel testo del provvedimento e tutti saremo più tranquilli.

al fatto che ci fosse una sicurezza anche per un'altra comunità. Non ho detto prima noi e poi loro, perché altrimenti non avremmo neanche ceduto la nostra motonave.

Come si sa, il provvedimento in esame dispone di cedere, come conseguenza di un accordo internazionale, a un altro Paese alcune unità navali.

Senatore Ferrari, ho fatto una riflessione rispetto alla sua segnalazione. Non solo nella relazione di accompagnamento, ma nello stesso articolo 1 si dice: «per incrementare la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno»; se il testo si fosse fermato qui, avrei potuto anche dire che c'è fondatezza in quello che lei ha testé citato. però anche: «nelle attività di controllo e di sicurezza rivolte al contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di essere umani, nonché nelle attività di soccorso in mare». Pertanto, con queste finalità, ritengo l'emendamento del relatore ammissibile. Invito

degli ultimi eventi di cui tutti siamo a conoscenza. Abbiamo voluto inserire, proprio per quello che diceva poc'anzi il Presidente sul tema della sicurezza e della salvaguardia in mare, in mare, un'adeguata preparazione in materia di primo soccorso e tutela dei diritti umani. Non si capisce allora perché si possa andare avanti con l'emendamento in cui si prevede di dotare delle unità navali nostre e, quindi, non oggetto del Memorandum internazionale sulla cui base noi oggi andiamo ad individuare il decreto-legge in cui cediamo dodici unità navali libiche, e invece per noi che chiediamo di rafforzare uno degli elementi qualificanti di quell'accordo e, cioè la formazione del personale libico in un scenario come quello che stiamo vivendo, non sia possibile non sia possibile inserire il rafforzamento del concetto del primo soccorso e della tutela dei diritti umani, che ha a che fare proprio con la salvaguarda della sicurezza in mare. Insistiamo quindi per votare a favore di questo emendamento.

rispetto alla concessione di unità navali alla Guardia costiera libica. Sono di pochi giorni fa le immagini del salvataggio di una donna - non lo diciamo in in ragione di una categoria di cui ormai si abusa nel commento della politica, cioè il buonismo, ma perché riportiamo la realtà dei fatti per come si sta configurando - Josefa, da parte della nave da parte della nave della ONG Proactiva Open Arms, aggrappata ai resti di un gommone in mare, in procinto di morire per ipotermia accanto ai cadaveri di un'altra donna e del suo bambino. Con il passare dei giorni, la ricostruzione di quanto avvenuto, testimoniata anche dalla presenza di un nostro deputato, l'onorevole Palazzotto, che è stato su quella nave, diventa sempre più chiara e conduce a una diretta responsabilità della della Guardia costiera libica, nonostante gli evidenti tentativi di manipolazione della realtà che hanno seguito le ore successive al salvataggio. Sembrerebbe, infatti, che la Guardia costiera libica, intervenuta per il recupero di 158 persone a bordo di un gommone, abbia abbandonato in mare le due donne e il bambino a causa del loro probabile rifiuto di interfacciarsi con un soggetto riconosciuto come pericoloso, la Guardia costiera libica, appunto. C'è poi da chiedersi in quale modo il gommone sia stato distrutto e se anche su questo profilo l'intervento della Guardia costiera della Libia sia stato determinante. Ricordiamo come lo scorso anno la ONG Proactiva abbia divulgato un video in cui venivano mostrati agenti della Guardia costiera libica sparare in aria per intimidire l'equipaggio di una delle due navi della ONG spagnola. Ecco, di fronte a tutto questo, di fronte alle immagini e alle denunce di organismi indipendenti come l'UNHCR o Amnesty International, che da mesi riportano le inaccettabili condizioni delle persone migranti in Libia, le violenze, le torture, gli stupri quotidiani, nonostante questo patrimonio di informazioni, i nostri Governi l'attuale, ma anche quelli che lo hanno preceduto - si ostinano a considerare la Libia come un interlocutore cui affidare la vita di centinaia di migliaia di persone. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità sarebbero più di 10.000 le persone individuate dalla Guardia costiera libica e rinchiuse in circa 20 centri di detenzione, e circa 662.000 i migranti, come riportato dal ministro Salvini qualche settimana fa durante un'informativa al Senato. Il nostro Governo vuol far passare il messaggio secondo cui la drammatica carenza di navi che consentono il salvataggio di migranti nel Mediterraneo possa essere risolta regalando unità navali alla Guardia costiera libica. Sappiamo bene, invece, come tale carenza sia da imputare principalmente alla decisione dei Governi europei, in primo luogo di quello italiano, di ostacolare il sistema di assistenza cui provvedevano proprio le organizzazioni non governative, ostacolando al contempo l'attivazione di canali di immigrazione regolari e di corridoi umanitari che consentano di salvare realmente la vita di migliaia di persone. evidente come il fine ultimo di questo Governo, che si muove in sostanziale continuità con le scelte dei Governi precedenti, forse è quello non di salvare

e urgenza che risulterebbe accettabile per un decreto-legge in materia di immigrazione, il salvataggio delle persone, non l'affidamento a soggetti che finora non hanno dimostrato alcuna attenzione non solo verso le norme internazionali ma nemmeno verso il più basilare rispetto di diritti umani. forse risuonare con maggiore impatto le parole del Segretario Generale dell'ONU anche in quest'Aula, il quale ha definito le condizioni dei migranti in Libia come crimini contro l'umanità. sembra pleonastico doverlo ricordare, ma, a quanto pare, non lo è - non ha un vero Governo, istituzioni stabili con cui interfacciarsi senza ambiguità; gran parte del territorio è infatti in mano a trafficanti di esseri umani, spesso in combutta con milizie, tribù e funzionari governativi. Lo Stato libico è totalmente depotenziato dai conflitti interni, con intere zone controllate da fazioni diverse che trattano direttamente con i trafficanti di esseri umani: non è chiara, dunque, la motivazione con cui ci apprestiamo ad affidargli la gestione di un fenomeno complesso come quello migratorio. La Libia - ricordiamo ancora - non riconosce nemmeno la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951. In questo contesto, ci sembra d'obbligo ricordare la decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che appena qualche mese fa ha sanzionato sei trafficanti di uomini libici, tra cui proprio l'*ex* capo della Guardia costiera al-Milad: i rapporti dell'ONU lo accusano infatti di "aver sparato sui barconi dei migranti per affondarli", aggredendoli in mare e vendendoli ai miliziani che controllano i centri di detenzione; un individuo che, al pari di questo Governo, ha mostrato una profonda avversione per le ONG, definite come braccio di servizi segreti stranieri. Con il provvedimento in esame ci sembra dunque di assecondare l'inaccettabile ricatto promosso dalle autorità libiche, che sembrano aver voluto questa è la nostra impressione - la disponibilità del nuovo Governo, così come di quelli che lo hanno preceduto, alla concessione di risorse e mezzi in cambio del blocco delle partenze. Ma questo - come sta dimostrando una lunga serie di *reportage* - sta facendo pagare il prezzo di questo braccio di ferro a centinaia di uomini, donne e bambini in palese contrasto con quanto affermato all'articolo 1 del decreto-legge in cui si parla di finalità di soccorso in mare; le unità fornite sono molto piccole: l'associazione Diritti e Frontiere ha segnalato, in tal senso, come le navi sembrino molto più indicate per intercettare e bloccare i barconi carichi di migranti sotto minaccia delle armi, piuttosto che per procedere a operazioni che garantiscano il salvataggio e il trasferimento verso un porto di sbarco sicuro. Proprio su quest'ultimo punto, inoltre, ricordiamo come l'ONU abbia dichiarato la Libia porto non sicuro ai sensi della Convenzione di Amburgo del 1979, un'affermazione confermata da recenti decisioni dei giudici di Ragusa Noi pensiamo che sia giusto votare contro questo provvedimento, che va esattamente nella direzione che ho descritto. E ci permettiamo di dire che, forse, bisognerebbe ripartire da alcune scelte che hanno caratterizzato il passato e che poi sono state drammaticamente e colpevolmente abbandonate. Penso a Mare Nostrum. Bisognerebbe ripartire dall'attivazione - come dicevo prima - di canali di immigrazione regolare ma, soprattutto, bisognerebbe ripartire dalla nostra umanità.

abbiamo sostenuto sin dal dibattito sul voto di fiducia che avremmo tenuto un atteggiamento da opposizione propositiva, che è qualcosa di più rispetto all'opposizione costruttiva che ci veniva chiesta. E lo stiamo dimostrando anche nei confronti del provvedimento in esame, un provvedimento che abbiamo discusso in maniera significativa nelle Commissioni per sopperire ad alcune carenze che erano emerse in merito al valore patrimoniale dei mezzi che venivano ceduti, alle coperture finanziarie, alle discrepanze, alle contraddizioni

ha risposto con una relazione tecnica molto esauriente che ha integrato - e in alcuni casi corretto - le note tecniche precedenti, tra l'altro sopperendo - per esempio - per quanto riguarda la valutazione del patrimonio, alla mancata stima. Quindi, abbiamo dato il nostro contributo affinché il provvedimento fosse fatto al meglio. Avremmo voluto fare di più, con gli emendamenti presentati prima in Commissione e poi in questa Assemblea, per rassicurare gli operatori della sicurezza (delle Capitanerie di porto e della Guardia di finanza) a cui vengono sottratti loro mezzi - in alcuni casi, gli esclusivi mezzi - senza avere la certezza che quegli stessi vengano sostituiti ove ve ne fosse la necessità.

i mezzi della Capitaneria di porto e della Guardia costiera. Riteniamo che anche questo sia un elemento aggiuntivo importante per meglio contrastare l'immigrazione clandestina e, eventualmente, soccorrere coloro che si trovassero in difficoltà nelle acque territoriali italiane o in quelle internazionali. Quindi, il nostro atteggiamento è di un'opposizione propositiva, tesa a migliorare i provvedimenti in questa sede o a contrastarli quando non li condividiamo, come - per esempio - sta accadendo con il decreto-legge disoccupazione, falsamente chiamato decreto-legge dignità, all'esame della Camera dei deputati. E questo è il nostro atteggiamento

Voglio, però, far notare che siffatto provvedimento oggi è inserito in un contesto politico di contrasto all'immigrazione ben diverso da quello che si è realizzato nel precedente Governo: un contrasto all'immigrazione che, soprattutto per impulso del Ministro dell'interno, sta vedendo il nostro Paese in prima fila in Europa, teso a svegliare tutti i Paesi affinché contrastino un fenomeno particolarmente grave che mette a repentaglio - lo ha sottolineato anche oggi, in questa sede,

le persone in questione, i migranti che fuggono dalla disperazione e dalla miseria, in qualche caso anche i profughi che fuggono dalla guerra, non fuggono dalla Libia; non fuggono dalla Libia; non sono libici. Fuggono da altre aree dell'Africa attraverso la Libia. Se il fenomeno si è creato, lo si è creato e lo si è ingigantito proprio perché la percezione che quelle popolazioni avevano, in Nigeria come in Corno d'Africa, era quella di una navigazione attraverso il Mediterraneo supportata poi dalle navi delle organizzazioni non governative. Mi ha colpito, cari colleghi, qualche anno fa la dichiarazione di alcune persone che portavano l'esempio molto semplice, e chiaro a tutti noi, secondo il quale qualunque pastore del Centro Africa,

le stesse conoscenze e informazioni sul mondo di cui venticinque anni fa era in possesso solo il Presidente della Repubblica americana.

è consapevole che esiste un mondo diverso e altresì che delle navi raccolgono i profughi nelle acque territoriali della Libia per poi portarli in Europa, quindi si muovono sulla base di questa illusione. Il telefonino trasmette siffatta speranza e centinaia di migliaia di persone, sulla base di quella immagine, spesso di quella illusione, finiscono in Libia nelle mani sanguinarie dei trafficanti di uomini, che sono peggiori dei trafficanti di droga. di droga. Questa illusione noi dobbiamo eliminare o se eliminiamo questa illusione e quelle immagini, noi freniamo alla fonte freniamo alla fonte la migrazione che parte dall'Africa centrale. Questo ci pone il problema anche di cosa fare per quei popoli e lo dico con grande responsabilità. Mi dispiace che nel dibattito molto politico, che si è aperto per alcune ore, nessuno abbia citato ad esempio,- come abbiamo già fatto in Commissione e in quest'Aula in altra sede e per pochi secondi il capitolo di pace che si è aperto nel Corno d'Africa. Lo sottolinea il Governo, lo sottolinea l'Europa e lo sottolinea questa Assemblea: se vogliamo fermare la migrazione biblica che viene da quelle terre e almeno un terzo dei migranti che cercano di giungere in Europa attraverso l'Italia parte da quelle terre - vorrei che il Governo, l'Italia e l'Unione europea cogliessero quei segnali di pace e di stabilizzazione che riguardano l'Etiopia, l'Eritrea, la Somalia citata in quest'Aula, il Sud Sudan e anche il Sudan e il Kenya, tutta un'area geografica particolarmente fondamentale per noi perché fonte del flusso di migrazione, talvolta di profughi che migrano

bloccare, per quanto ci riguarda, la migrazione clandestina che sbarca nei porti italiani; dall'altra parte, certamente con questo provvedimento, che non è piccolo, perché non si limita a fornire dodici navi all'autorità libica, dà un segnale importante all'autorità libica di legittimazione di quelle istituzioni, e le istituzioni libiche hanno bisogno di essere legittimate; e dà il segnale importante all'Unione europea

dalla sudditanza monetaria alla Francia ed era una minaccia per tutti i Paesi del Centro Africa che subiscono siffatta dominazione. Io Io credo che questo segnale sia molto più importante delle dodici motovedette concesse alle autorità libiche: è un segnale alle istituzioni libiche, è un segnale all'Unione europea,

al nostro esame è un provvedimento certamente limitato e relativamente semplice dal punto di vista tecnico. È però evidente che si inserisce in un contesto geopolitico difficile e complesso,

leggero. In queste scelte, infatti, si mescolano ragionamenti e valutazioni di tipo politico, diplomatico, a volte economico e commerciale, che si mischiano con questioni che hanno a che fare con la sfera etica, con i convincimenti personali, con i principi e i valori alla base della nostra cultura. Ed è evidente che, quando ci si confronta con contesti diversi, esse creano anche conflitti identitari. complicato e difficile maturare queste scelte. Siamo consapevoli anche noi - come ha sottolineato la senatrice Bonino nel suo intervento della situazione maledettamente complicata in Libia, di una statualità che non esiste, ma che non esiste oggi così come non esisteva prima. Era originale infatti anche la statualità ai tempi del *rais*, quando le diverse tribù - le stesse tribù che adesso si organizzano in maniera diversa - erano unificate in una sorta di sistema feudale, dove egli era il feudatario e i capi tribù erano i vassalli e i valvassori: già allora c'era un meccanismo di scambio. stesso vale anche per il concetto stesso di diritti umani e per la concezione di dignità umana, che là è diversa. Dunque, per questo motivo, non dovremmo avere rapporti e non dovremmo tentare di costruire dei ponti con un Paese che è di fronte a noi, la cui relazione è strategica, non fosse altro per il fatto che siamo immersi nel Mediterraneo e, anche non volendo, subiamo gli effetti negativi di un contesto non stabilizzato? Penso che dobbiamo tornare indietro. È stato citato più volte il Trattato di Bengasi. La verità è che il vero spartiacque è stata è stata l'intuizione di Romano Prodi nel 1997: lì sì che sono cambiati i rapporti con la Libia. Per anni ci fu quasi un embargo, anzi un vero e proprio embargo nei confronti di quello che quello che gli Stati Uniti definivano un *rogue State*, con il quale non dovevamo avere rapporti, tanto che c'erano sanzioni unilaterali degli Stati Uniti e sanzioni multilaterali del sistema delle Nazioni Unite. Prodi, prima da Presidente del Consiglio e poi da Presidente della Commissione europea, fu di portare quello Stato, che poteva diventare la palestra del terrorismo islamico, il luogo in cui cresceva la proliferazione di armi di distruzione di massa, dentro un dialogo multilaterale, provando a risolvere anche problemi commerciali ed economici, che da anni gli italiani e le nostre stesse imprese chiedevano di risolvere. Diplomazia economica, politica, capacità di riportare la Libia dentro la comunità internazionale e di superare l'episodio tragico di Lockerbie: fu quella l'intuizione vincente. Su quella scia si innestò anche la diplomazia di Berlusconi, certamente con un'impronta più economica. L'errore fu il dissennato intervento in Libia. Pedagogicamente e didatticamente si potrebbe spiegare alla senatrice che è intervenuta prima che esso fu appoggiato dal Governo di centrodestra. Noi allora eravamo all'opposizione ed è bene magari ogni tanto ricordare anche questi passaggi. Poi fu difficile portare avanti questo tipo di lavoro, che fu ripreso dai Governi di centrosinistra, in particolare con il Memorandum Gentiloni Silveri, firmato il 2 febbraio del 2017. Ecco, lì dentro c'è una strategia complessiva

interventi di cooperazione e di aiuto a quelle comunità che pagano un prezzo altissimo alla tratta di esseri umani. Qui ci soffermiamo solo sulla parte finale, sul pattugliamento delle coste, sull'intervento nel Mediterraneo, ma non sulla cooperazione allo sviluppo e non su una collaborazione per sigillare i confini sud della Libia, che sono maledettamente difficili, perché c'è il deserto. E ricordo ancora una volta che, quando noi abbiamo proposto la missione in Niger, chi oggi sta sui banchi della maggioranza votò contro, mentre al contrario bisognava dare il segnale quello era il primo momento in cui si affrontava anche il tema della tratta degli esseri umani. Vi è poi la condizione precaria in cui si trovano i centri permanenti in Libia. in Libia. Nell'ordine del giorno G1.100 - e mi dispiace che abbiano votato contro il nostro emendamento - noi abbiamo chiesto anche un'attenzione alla collaborazione con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni e con l'Alto commissariato per i rifugiati, decisivo perché non solo il centro che sta costruendo l'UNHCR ma anche gli altri gestiti dai libici abbiano un controllo delle organizzazioni internazionali, per alzare lo *standard* e il livello minimo dei diritti umani. È a tal riguardo che manca l'approccio di questo Governo. Diamo le motovedette, e va bene, ci siamo. Tuttavia, nel momento in cui si danno le motovedette, chiediamo che in tutti i centri ci siano anche i rappresentanti delle organizzazioni internazionali legate alle Nazioni Unite. È così che si fa, è una regola semplice. La diplomazia prevede questo: motovedette, ma anche la capacità di innalzare il livello dei diritti umani, la capacità di costruire istituzioni democratiche. È questo il motivo per cui noi voteremo a favore del provvedimento in esame, ma non saremo più disposti in futuro - come abbiamo scritto nel nostro ordine del giorno e nell'emendamento - ad approvare ulteriori provvedimenti che si limitino solo al contrasto dell'immigrazione nel Mediterraneo e non affrontino i temi centrali di come affossare la tratta degli esseri umani, controllare i confini del Sud della Libia e attuare un grande piano complessivo di aiuti alla cooperazione allo sviluppo. Solo se faremo così vinceremo la nostra battaglia in Libia. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi senatori, il nostro Gruppo voterà convintamente a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2018 per almeno tre ordini di ragioni che mi accingo a declinare: sotto il profilo della coerenza programmatica, della ricostruzione di una linea chiara di relazioni internazionali, diplomazia e politica estera del Paese nel quadrante Mediterraneo e non solo, dell'interesse nazionale a ristabilire il ruolo di *partner* principale politico della Libia nella sua interezza. Il contratto di Governo, su impulso determinante della Lega di Matteo Salvini, ha posto con fermezza l'esigenza di affrontare la gestione dei flussi migratori clandestini con una prospettiva nuova

unitamente ai meccanismi poco trasparenti previsti per la loro gestione, hanno costituito un elemento sicuramente attrattivo per la criminalità organizzata. Non è civilmente né tantomeno umanamente tollerabile assistere passivamente all'azione criminale di scafisti che quotidianamente alimentano una vera e propria tratta, lucrando sulla pelle dei migranti e seminando disordine e morte nei nostri mari. Per andare alla radice del problema, non si può prescindere da una strategia condivisa con la Libia, che in questi anni è stata scelleratamente sprofondata nel caos dall'improvvida decisione di bombardare e destituire il regime al potere senza una seria e concreta alternativa unitaria divenendo così il principale collettore di questi fenomeni. Osservatori indipendenti accreditati hanno stimato che oramai il *business* del traffico migratorio rappresenta il 30 per dal quale sempre più ampie porzioni della società libica traggono sostentamento, con il rischio reale che questo modello di economia illegale diventi strutturale e difficilmente riconvertibile in quei territori. Oggi il nostro impegno deve essere il supporto alle ricostituite autorità libiche per sviluppare un'efficace politica di difesa delle proprie frontiere a Sud, specialmente mediante accordi bilaterali con i Paesi centroafricani e del Sahel, ma soprattutto un controllo puntuale del proprio confine lungo la costa settentrionale che guarda all'Italia. Attualmente la Guardia costiera libica dispone di appena quattro motovedette piuttosto vetuste e operativamente limitate, sia sotto il profilo delle dotazioni di bordo che di personale, dismesse a suo tempo della Guardia di finanza italiana e successivamente donate dai Governi Berlusconi e Gentiloni Silveri nell'ambito dei numerosi accordi bilaterali di cooperazione sottoscritti tra i due Paesi. In questa cornice si inserisce il provvedimento in trattazione che, nel solco della collaborazione bilaterale, si pone sul piano della concretezza dell'azione offrendo alle autorità libiche una flotta che va a quadruplicare l'attuale disponibilità di unità navali e, dunque, degli addetti al pattugliamento e al controllo delle acque territoriali, unitamente alla indispensabile attività addestrativa e di formazione del personale degli organi per la sicurezza costiera. Queste misure concorrono, per altro verso, a dare effettività all'azione del Governo libico. Infatti, non appare realistica una soluzione complessiva dei molteplici problemi connessi all'attuale condizione del territorio libico senza un consolidamento del Governo di al-Sarraj che lo elevi a uno *status* compiuto, emancipato dalla percezione di ente fiduciario della comunità internazionale. che la collega Bonino sia assente ora dall'Aula. Noi sappiamo bene quale sia la fondazione della Libia, ma lei non può fingere di non sapere perché è così e chi ha destabilizzato il Paese. Quel Paese è stato destabilizzato dalle scelte e dagli interessi di gruppi di potere internazionali coi quali voi avete consuetudine di rapporti, Se l'ex provincia ottomana del Fezzan è segnata dalla lotta tra le minoranze tuareg, i tebu e le tribù arabe come gli awlad suleiman, forse c'è una relazione con le politiche dell'amministrazione Obama, finalizzate a favorire la nascita di Governi tribali e islamisti. Oggi noi seguiamo la linea della legittimità internazionale dialogando con l'unico interlocutore riconosciuto. Lei, senatrice Bonino, si è detta legalitaria, ma temo che stia declinando questo concetto nel senso di legalizzare ciò che legale non è, cominciando a praticarlo anche prima che lo diventi. I suoi canali legali di ingresso a chi sarebbero rivolti, a quanti e con quali requisiti? Già esistono forme legali per entrare nel Paese, ma qui stiamo parlando di immigrazione clandestina e quindi illegale. *(Applausi Dal mio Gruppo può essere stata contestata per questo, ma mai è giunta da questi banchi un'offesa, mai una minaccia o un insulto: non è un modo che ci appartiene. *(Applausi Quale sarebbe l'alternativa? L'alternativa a non dialogare con al-Sarraj è il rischio esiziale che, sotto la spinta delle diverse forze insurrezionali ivi operanti, si giunga alla definitiva dissoluzione di uno Stato libico. Il Consiglio di sicurezza ha sempre espresso risoluzioni per l'unità della Libia e contro ogni ipotesi di secessione. Ma, se la situazione dovesse precipitare, non vi sarebbero grandi margini di recupero. Sotto un ulteriore profilo, con questo provvedimento auspichiamo che il Governo riprenda complessivamente e con una più ampia prospettiva il ruolo di iniziativa politica e diplomatica che il Paese aveva smarrito negli anni, soprattutto riguardo alla Libia. Da troppo tempo, infatti, l'Italia ha rinunciato al proprio ruolo naturale di *leader* di riferimento per la regione, accettando supinamente che la Francia guadagnasse talmente terreno da porsi, a maggio di quest'anno, come unico e privilegiato mediatore tra le diverse fazioni in conflitto, nella chiara ricerca di aprire un nuovo mercato per gli interessi francesi, nuove commesse per le proprie aziende e per l'industria bellica d'Oltralpe. Per parte nostra, invece, dobbiamo tutelare la presenza - ad esempio - dell'ENI sulla sponda mediterranea dell'Africa, difendendo gli investimenti fatti negli anni per la ricerca di giacimenti di gas e petrolio, ai quali punta con forza la Total Elf. Ciò significa restituire senso e dignità al concetto di interesse nazionale, troppo spesso obnubilato dall'esigenza di assecondare scelte ideologiche globaliste e *radical chic*. *(Applausi dai Per tutte queste ragioni, confermando il voto favorevole del Gruppo, auspichiamo un'analoga espressione da tutto il Senato.

lungimirante, razionale, solidale, ferma e responsabile, ce lo impone. Vorrei chiarire immediatamente un punto. Ho detto solidale perché siamo stati un grande Paese e nel nostro programma c'è anzitutto la difesa della vita di coloro che si lanciano in mare nella speranza di trovare non solamente approdi sicuri, ma anche un tipo di vita diverso. Difendere la vita significa effettuare operazioni di salvataggio. Tuttavia, siamo al tempo stesso fermi nel comprendere che la situazione reale dell'Italia - e noi dobbiamo confrontarci con il mondo reale non è tale da consentire l'arrivo di chicchessia, di tutti coloro che avrebbero il desiderio di partire dall'Africa per venire in Italia. Sappiamo che l'Africa ha 1.200 milioni di abitanti. un continente immenso. L'Austria ha chiuso i suoi confini e la Francia ha fatto la stessa cosa. I confini degli Stati non sono cessati; la politica internazionale non ha decretato la cessazione dei confini dell'Italia. Per questo motivo, riteniamo che il primo fronte di intervento per le operazioni sia umanitarie che di contrasto all'immigrazione clandestina debba essere proprio a ridosso delle coste libiche, nel Mediterraneo. Questo è il nostro intendimento.

la preparazione delle marinerie libiche e, soprattutto, di quelle imbarcazioni, con l'auspicio che possano entrare in servizio in tempi rapidi. Credo che questo sia il regalo più bello che possiamo fare non solamente alla Libia, ma all'Italia e all'Europa e - mi permetto di dire - anche a quegli immigrati che sperano di arrivare, ma che non si rendono conto delle tragedie che hanno trasformato il Mediterraneo in un grande cimitero. Ci sono 30.000 morti che Gruppo FI-BP)*. E ciò è avvenuto per scellerate politiche di accoglienza, perché si è raccontato che qui si poteva fare di tutto.

Deve esserci un vero e proprio piano Marshall per l'Africa. Dobbiamo investire in quelle terre con l'aiuto e l'intervento anche di altre nazioni. Dobbiamo sicuramente presidiare il confine sud della Libia. Dobbiamo cominciare a pensare anche noi - lo avevamo indicato nel nostro programma - a un pattugliamento dell'area Sud del Mediterraneo, con un blocco navale per disincentivare le partenze. A questo punto mi chiedo, in effetti, dove è l'Organizzazione delle Nazioni Unite e che cosa ha fatto per l'Africa negli ultimi anni? Come mai ci siamo ridotti in queste condizioni? Realizziamo, laddove possibile, con investimenti, degli *hotspot* al confine Sud della Libia.

È chiaro che non lo posso chiedere a colui che fa la traversata. È necessario quindi aprire questi *hotspot*, rafforzare la nostra ambasciata in Libia, riuscire a normalizzare la realtà libica.

signor Presidente, riteniamo che questa operazione debba essere solo l'inizio di un grande progetto per l'Africa, un grande progetto di protezione anche per la nostra Nazione. Mi limito a ricordare che è stato approvato e accolto anche dal Governo un ordine del giorno molto importante, che va nella direzione di aiutare gli imprenditori, le nostre imprese, le 100 imprese che ho citato anche in discussione generale.

importante, ma semplice e, nella sua perimetrazione politica, parla di qualcosa di veramente specifico, di dodici motovedette che noi stiamo fornendo, dopo una

altrimenti in quello che a me piace definire contro populismo; voi ci accusate di essere dei populisti, ma probabilmente è peggio il contropopulismo, cioè dire sempre ed ostinatamente delle falsità nella

è veramente difficile fornire questi oggetti a un Governo che non esiste, ad uno Stato che non esiste. Dobbiamo anche essere obiettivi, perché quando si tratta di rapporti commerciali, quando si parla di fare *export* in Paesi che sono completamente destabilizzati, guarda caso, l'interlocutore siete riusciti a trovarlo sempre. Allora probabilmente dovremmo fare uno sforzo e riuscire a trovarlo anche in questi ambiti. Gli obiettivi di questo decreto-legge erano tre sostanzialmente: il controllo dei flussi migratori, un un tentativo di stabilizzare la Libia e, ripeto, il contrasto al traffico di esseri umani. Anche su questo va chiarito un punto. In passato c'è stata raccontata una Libia che in realtà non esisteva. Quando il segretario generale della NATO Stoltenberg veniva qui in Senato a raccontarci

una Tripoli stabile politicamente mentre contemporaneamente Stoltenberg ci parlava di una Tripoli in cui c'erano 87 fazioni in combattimento, cioè una dietro ogni angolo.

Il nostro ministro Moavero Milanesi ha detto che alcuni di quei Trattati, che sono sostanzialmente congelati, vanno riaperti per un giusto dialogo con un Paese che è vicino a noi, che è sostanzialmente confinante perché è il primo Paese che troviamo al di sotto del nostro mare. Ma c'è un altro punto importante che ci spinge a votare a favore di questo provvedimento. Nel corso della discussione e anche nei contenuti della relazione, sono emerse delle criticità. Proprio ad avvalorare il fatto che non c'è continuità con il passato, lo stesso Governo, nella persona del sottosegretario Molteni, che ringrazio per il suo lavoro,

è un ulteriore segnale di discontinuità con il passato ed è sicuramente una nota nuova, una nota unica.

Uno dei problemi di quelle aree è che sono state per molti anni governate da entità anche dittatoriali. Addirittura molti anni fa c'era il faraone. Fortunatamente il faraone ora non c'è più. Ce n'è qualcuno ancora in giro e purtroppo ce lo teniamo.

per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale»,

di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità da parte del comune di Bari degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari. Il testo all'esame non è stato oggetto di modifica da parte della Commissione giustizia. Nessuno degli emendamenti presentati, infatti, è stato approvato. Nel corso della discussione non sono mancati rilievi critici sul provvedimento, il cui contenuto tenterò di riassumere nella illustrazione che mi appresto a svolgere. Nel merito il decreto-legge in conversione consta di tre articoli. L'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari e del corso della prescrizione. Per i procedimenti penali pendenti (il provvedimento non chiarisce espressamente a quale data tali procedimenti debbano risultare pendenti, ma per questa ragione sarà presentato un ordine del giorno *ad hoc* che mi riservo di illustrare meglio nel prosieguo) il decreto-legge sospende i termini di durata delle indagini preliminari; i termini previsti dal codice processuale penale, a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni. Si tratta di sospensioni che, a differenza di quanto denunciato da alcuni colleghi dell'opposizione, non minano affatto il diritto alla difesa; anzi, per larga parte ne sono a garanzia. Parliamo peraltro di una sospensione che non opera per tutti i procedimenti. A ben vedere, infatti, il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni. In particolare, la sospensione non opera per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo, nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare. Tale sospensione, inoltre, non opera con riguardo ai processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare personale, in presenza di profili di urgenza valutati dal giudice procedente. Quest'ultima previsione - mi permetto di ricordare - è stata inserita dalla Camera nel corso dell'esame in sede di conversione e non è stata modificata dalla Commissione giustizia del Senato. L'articolo 2 del decreto-legge reca, poi, la clausola di invarianza finanziaria, che ritengo opportuno leggervi testualmente: «Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». Mi pare evidente che tale articolo fughi ogni dubbio circa la presunta eccessiva onerosità delle misure contenute nel decreto-legge in conversione. In merito alla congruità della clausola d'invarianza finanziaria, mi permetto di segnalare all'Assemblea che, proprio nella giornata di ieri, si è espressa favorevolmente - approvando un parere non ostativo sul testo del decreto-legge - anche la Commissione bilancio. L'articolo 3 contiene infine la norma relativa all'entrata in vigore. Prima di concludere il mio intervento, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni su una questione particolarmente discussa sia alla Camera sia al Senato. Vorrei precisare, per conto di tutti, che l'individuazione dell'immobile da destinare alla nuova sede del tribunale pugliese è una questione che esula completamente dal decreto-legge in conversione. Il provvedimento - lo ribadisco - si propone di affrontare responsabilmente danni che altri hanno compiuto negli anni e, e, attraverso la misura straordinaria della sospensione, che, come ribadisco, opera per un lasso di tempo estremamente limitato - stiamo parlando di tre mesi - fronteggia mesi - fronteggia una situazione emergenziale, che vede impossibile lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nella città di Bari.

ha dominato parte della cronaca di queste settimane, e vale la pena riepilogarla: la condizione fortemente critica degli edifici del tribunale e della procura di Bari, la dichiarazione di inagibilità

distaccata del tribunale di Modugno, le tensostrutture, che tanta discussione hanno legittimamente prodotto. Infine, il provvedimento oggetto di questa discussione, sospende i termini stabiliti dal codice di procedura penale per la durata della fase delle indagini preliminari e della relativa udienza preliminare, i termini in materia di inammissibilità e decadenza e quelli fissati per la proposizione di impugnazione o reclami fino al 30 settembre 2018, come ricorda il relatore. In qualità di membro della Commissione bilancio, Presidente, vorrei intervenire in merito ai profili finanziari di questo provvedimento, alla quantificazione degli oneri e alla copertura dei medesimi. Il Governo al Ministero della giustizia ha depositato, su richiesta del relatore in Commissione bilancio, un aggiornamento della relazione tecnica che specifica, come richiesto dal relatore stesso, alcuni elementi informativi in merito alla possibile quantificazione degli oneri relativamente ad un aspetto particolare, cioè la notifica degli atti penali

ad un'altra cosa: avrebbe un costo molto superiore quantificato in 11 euro a notifica. Sulla base di queste stime, il Ministero quantifica in 60.000 euro il costo complessivo delle notifiche non telematiche, un onere, secondo il Ministero, che può essere coperto sostanzialmente dai risparmi sulle spese di giustizia derivanti dalla temporanea sospensione delle attività processuali negli uffici giudiziari di Bari e, nel caso in cui questi risparmi non fossero sufficienti, comunque attingendo al capitolo 1550 (Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari). Queste stime e queste valutazioni noi le abbiamo contestate in sede di Commissione bilancio e torniamo a contestarle Contestiamo la quantificazione degli oneri di questo provvedimento, perché ci sembra non realistica la stima del 90 per cento delle notifiche effettuate per via telematica. È vero che nel rapporto con gli avvocati ormai tutto avviene secondo procedure telematiche, ma molte di queste notifiche devono essere fatte agli imputati e, nella stragrande maggioranza dei casi, gli imputati non hanno posta elettronica certificata per cui le notifiche vanno fatte secondo posta ordinaria o a mano, con un costo - come ricordavo in precedenza - di 11 euro a notifica. Noi, quindi, riteniamo che i costi rischino di essere notevolmente superiori rispetto alla stima di 60.000 euro fatta dal Ministero della giustizia e portata in Commissione bilancio del Senato, riteniamo che vi sia il concreto rischio che i risparmi derivanti dalla sospensione dell'attività del tribunale non siano affatto sufficienti a coprire questi oneri, che potrebbero essere molto superiori ai 60.000 euro e riteniamo che rischino di compromettere la clausola di invarianza finanziaria che, come ricordava il relatore, sostiene che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che questi oneri debbano essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ricordo, però, che lo stesso capitolo 1550 («Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari») si riferisce alle spese

sono state utilizzate per giudicare il decreto-legge in questione, quello che avrebbe dovuto avere parte decisiva per risolvere la questione del tribunale di Bari: fallimentare, irragionevole, incompetente, in malafede, una mostruosità e, per concludere, incostituzionale. È evidente, quindi, che tali giudizi unanimi, la maggior parte dei quali provenienti da giuristi addetti ai lavori, non possono essere certo ascritti a una rivalità politica o a consueta dialettica tra maggioranza e opposizione. Si tratta, infatti, di obiezioni tecniche e severe prese di posizione indicative di una criticità, sostanziale e formale, che il Governo non può ignorare e che abbiamo il dovere, in sede di conversione del decreto-legge, di valutare nell'interesse particolare della situazione oggetto del provvedimento, ma soprattutto nell'interesse generale di alcuni principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, che non possono essere bypassati a cuor leggero, senza tener conto delle conseguenze disastrose per la realtà giudiziaria. Infatti, Forza Italia ha presentato questa mattina una pregiudiziale di costituzionalità, che è stata ahimè respinta a maggioranza dall'Assemblea, poiché, qualora il decreto-legge venisse convertito, le conseguenze delle eccezioni di costituzionalità, che verranno sicuramente sollevate nel corso dei processi, saranno incalcolabili. Il ministro della giustizia Bonafede, incontrando ai primi di giugno avvocati, magistrati e personale del tribunale barese, aveva assicurato una soluzione rapida per ripristinare le condizioni di sicurezza per gli operatori della giustizia e riavviare tutti i servizi all'utenza: il risultato è stato diametralmente opposto, al punto che le camere penali di Bari affermano oggi di preferire i processi nella tendopoli in piena estate, con i disagi già sperimentati nelle scorse settimane, rispetto alla sospensione dei termini.

ma si tratta comunque di elementi di valutazione, che incidono sul giudizio negativo complessivo, che purtroppo l'intera vicenda suscita, frutto di superficialità o anche di scarsa conoscenza del territorio. Di fatto, purtroppo, il rischio di complicare una situazione già gravissima è palese. Bisogna comunque, a onor del vero, riconoscere che l'attuale dramma del tribunale di Bari ha radici sicuramente risalenti nel tempo, trattandosi di una situazione già nota da moltissimi anni, ma purtroppo ignorata dalle amministrazioni locali del tempo (il sindaco Emiliano in testa), fino al prevedibile collasso degli ultimi mesi. Addossare però responsabilità pregresse sarebbe solo un mero esercizio di stile e quindi, come tale, inutile. La vicenda è senza dubbio complessa, per cui tanto più inadeguata appare oggi la soluzione semplicistica proposta, sia dal punto di vista giuridico, attraverso la sospensione dei termini processuali, che dal punto di vista logistico, con la scelta appunto dell'edificio provvisorio che deve ospitare le aule giudiziarie. Bisogna purtroppo riconoscere che, anche in questo caso, l'approccio del Governo appare in linea con una generalizzata tendenza ad offrire soluzioni semplici a problemi complessi; soluzioni che, chiaramente, non tardano a rivelarsi inadeguate, manifestando tutta la loro debolezza. Ciò sarebbe anche il male minore, se non fosse che intervenire con un provvedimento inadatto in una materia dalle innumerevoli implicazioni e ripercussioni sulle realtà professionali di tantissimi operatori del diritto e sulle vite di tantissimi cittadini, già penalizzati dai tempi biblici della giustizia italiana, comporta una pluralità di ricadute negative, che rischiano di aggravare *sine die* la situazione generale, piuttosto che risolverla. Dopo i mesi di sospensione sarà infatti necessario notificare migliaia di avvisi alle parti e ai difensori per fissare nuovamente le udienze, paralizzando a tempo indeterminato i processi. Soprattutto, il Ministro dovrebbe spiegare perché questa pseudo-emergenza, che reale emergenza non è, poiché ampiamente prevista, giustifica la sospensione dei diritti dei cittadini, ma non procedure d'urgenza e finanziamenti straordinari. I numeri confermano il *caos*: si parla di circa 72.000 procedimenti per almeno 100.000 notifiche: a quale costo? Il Ministero dice soltanto 60.000 euro, ma assolutamente esprimo i miei forti dubbi. Per farlo gli uffici impiegheranno mesi, se non anni, e intanto la prescrizione comincerà di nuovo a correre. Quale è il senso, dunque, di questa sospensione, nel quadro generale della situazione giudiziaria? Forza Italia rifiuta la soluzione temporanea, parziale e incostituzionale contenuta nel decreto-legge e indica invece la via della procedura d'urgenza, attraverso una norma che conferisca allo stesso Ministro poteri straordinari, in modo da poter derogare ai vincoli urbanistici e procedere al trasloco nell'immobile definitivo che sarà ritenuto idoneo. Se di reale emergenza si tratta, tratta, si abbia il coraggio di affrontarla con gli strumenti più incisivi a disposizione, piuttosto che ricorrere a rimedi di basso cabotaggio, apparentemente risolutivi, ma dagli effetti disastrosi nel lungo termine. A tutto questo non ci stiamo, nell'esclusivo interesse dei cittadini.

peraltro, in un quadro politico dove residua, in modo sempre più evidente ed imbarazzante, quella che mi viene spontaneo definire come schizofrenia.

Dapprima, infatti, abbiamo avuto una furia cieca, ossessa, che ha spinto il Ministro della giustizia a emanare con urgenza il decreto-legge una furia che paga subito il suo limite, dal momento che le condizioni riportate in premessa del decreto-legge e a giustificazione della sua necessità ed urgenza oggi non sussistono più: le tende sono state smontate. Allo stesso tempo, stiamo assistendo ad una vera e propria ritirata, ad una eclissi del ministro Bonafede; una eclissi solo parziale perché se da un lato continua a dimostrare, anche con l'assenza di questi giorni, il suo non voler continuare a metterci la faccia su questa vicenda, lo stesso non può dirsi per il provvedimento che per questioni meramente numeriche purtroppo sarà comunque verbis*, la congiunzione astrale di questo inizio legislatura sta inficiando negativamente il rapporto tra il MoVimento 5 Stelle e la decretazione d'urgenza;

Tale difficoltà si ritrova già nel titolo di questo provvedimento, dal momento che il ministro Bonafede ha deciso di conferire nuovo significato alla parola «svolgimento» dei procedimenti e processi penali, perché a Bari la giustizia è stata di fatto sospesa, bloccata, senza avere, però, la conseguente capacità di portare a fondo questa scelta drastica per gestire, così, in modo maturo e responsabile, gli effetti scaturenti da tale determinazione. Per questo, in mille modi abbiamo chiesto al Guardasigilli di assumere il ruolo di commissario straordinario; lo abbiamo chiesto noi e lo hanno fatto in tanti, soprattutto tra gli operatori. una scelta forte, forse l'unica capace di calmierare la forza degli effetti negativi del decreto-legge da lui voluto.

cancella diritti costituzionali, annacqua procedimenti, affoga distinzioni di rilievo, come quella tra istituto sostanziale e processuale della prescrizione; serve aceto alla bocca di quegli avvocati ai quali avete deciso di non sospendere i termini di scadenza delle rate degli oneri previdenziali e di quelli fiscali. Tutto questo per non ingarbugliare ulteriormente le acque con la clausola dell'invarianza finanziaria, ma - sia ben chiaro - va chiarito chi pagherà le notifiche, dal momento che continuiamo a credere come impossibile la copertura tramite posta elettronica di almeno 60.000 notificazioni. Ciò che più duole e rammarica nel commento al provvedimento in discussione è la cocciutaggine, la chiusura totale al confronto che ha avuto il ministro Bonafede. È riuscito in un'opera titanica di ricomposizione di un fronte storicamente molto frastagliato. È riuscito a compattare, scontentandoli, magistrati, avvocati, amministrativi del tribunale di Bari: tutti concordi nel contestare aspramente il decreto-legge ed i relativi contenuti. Possibile che tutti sbagliano? Possibile che non vi sia venuto il dubbio che forse l'atto in esame oggi è perfettibile, come da sempre si insegna? È possibile che non c'era spazio per accogliere anche qualche minima levigatura, lasciando così indicativamente aperta da parte del Governo la disponibilità al confronto e alla dialettica? La risposta è tanto semplice quanto perentoria: un secco «no». Il ministro Bonafede ha preferito semmai anticipare, in modo preoccupante e distopico, la concezione che il MoVimento 5 Stelle sembra nutrire del Parlamento, dei suoi nobili luoghi e dei suoi autorevoli rappresentanti, e che il CEO, Casaleggio, ha vaticinato in un'intervista di un paio di giorni fa. Al confronto schietto e diretto con i rappresentanti votati dal popolo in modo democratico, egli ha preferito la comunicazione monodirezionale della diretta Facebook, salvo poi capitolare tornare a Canossa di fronte alle preoccupanti ombre che incombono sull'individuazione della nuova sede del tribunale di Bari. Nel mancato ripensamento e quindi correzione di rotta,

a qualsiasi permeabilità volta alla ricerca di una saggia sintesi, e non invece l'ostinata chiusura in un fazioso oltranzismo, inopportuno e dannoso.

la questione del Palagiustizia di Bari affonda le proprie radici, non come è stato detto qualche minuto fa, nel 2010, ma nel lontano 2005, quando l'allora sindaco impedì di fatto la realizzazione del progetto della ditta Pizzarotti di Parma, di realizzare un polo unico della giustizia, quello che la città di Bari voleva già tempo. In quel progetto, vincitore di una ricerca di mercato, vi sarebbe stata certamente la soluzione all'annosa questione dell'edilizia giudiziaria a Bari. Essa avrebbe evitato, inoltre, il verificarsi dell'assurdo ed ignobile quadro delineatosi in questi giorni. Infatti, è tristemente noto a tutti che, a seguito dell'indagine tecnica affidata dal procuratore della Repubblica di Bari, dottor Giuseppe Volpe, all'ingegner Vitone, il cui esito si traduceva nel potenziale pericolo di crollo della struttura ove veniva amministrata la giustizia penale a Bari, seguiva la sospensione dell'agibilità del palazzo, a firma del sindaco Decaro. Così, tra l'incredulità e la piena emergenza, il 26 maggio venivano montate nel parcheggio sterrato dinanzi al tribunale tre tende con bagni chimici all'esterno, per consentire, in un'atmosfera surreale, la formale celebrazione delle udienze in calendario, al sol fine di disporre il rinvio di tutti i processi penali ordinari; un rinvio concesso senza una visione del futuro e solo per tamponare l'emergenza.

Questa situazione drammatica si è protratta per quasi un mese, dal 28 maggio al 22 giugno, durante il quale magistrati, cancellieri ed avvocati sono stati costretti ad esercitare il proprio lavoro in condizioni indegne ed indecorose, ben lontane dall'idea di un Paese civile. A porre fine a questa pagliacciata (perché, signori, di pagliacciata si è trattato), il decreto-legge del Governo che ha sospeso l'attività penale ordinaria nel capoluogo pugliese sino al 30 settembre prossimo. Così, a distanza di un mese, dal 1° luglio 2018, è stata smantellata la tendopoli nel parcheggio sterrato del Palagiustizia di Bari, ma purtroppo ciò non ha affatto risolto alcun problema. Non bisogna sottacere che la permanenza per oltre dodici anni degli uffici giudiziari all'interno dello stabile a rischio crollo, ben nota alle forze politiche di governo a livello sia locale, che nazionale, va senza dubbio alcuno ricondotta nella miope azione di chi ha ostacolato in ogni modo la la realizzazione del progetto Pizzarotti. Quei signori hanno costretto gli operatori del diritto a esercitare la giustizia e i cittadini a fruirne in un palazzo dichiarato abusivo sin dal 2005, del quale erano note le gravi problematiche strutturali, con la promessa che sarebbe stata una soluzione temporanea: per poco tempo - dicevano - giusto quello che serve per trovare un'alternativa valida e definitiva. Bene, miei cari signori, da allora sono passati ben dodici lunghi anni. Ebbene, le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e si traducono nel più assoluto svilimento dell'immagine della giustizia, nella svilente considerazione che nel capoluogo pugliese la giustizia penale, tra i capisaldi di ogni democrazia, è negata. Di fatto, non solo l'azione di questo qualcuno non è stata volta alla risoluzione della problematica relativa all'edilizia giudiziaria, ma anzi è stata causa determinante di quanto sta ancora accadendo a Bari. Per rimediare agli errori, imperdonabili, commessi in passato, sono necessarie delle misure importanti, non ultima la presa di coscienza che la soluzione alla questione edilizia giudiziaria la si può rinvenire solo in un intervento serio e importante. Non è più tempo di trasferimenti temporanei che poi diventano soluzioni definitive, come accaduto in passato. dicasi per la sospensione della prescrizione prevista dal decreto-legge emanato dal Governo per fronteggiare l'emergenza. Questa, signori miei, non è la soluzione al problema del Palagiustizia, ma anzi significa scaricare sui cittadini (indagato e imputato) gli evidenti errori della politica. Al centro di tutto - e qui mi rivolgo alla maggioranza - avrebbero infatti dovuto esserci loro, i cittadini indagati o imputati, che sono indagati e messi sotto processo pur essendo assolutamente innocenti o che, comunque, attendono di vedere definita la propria posizione. È a queste persone che abbiamo il dovere di dare delle risposte concrete, che non si possono tradurre nell'ulteriore dilatazione dei tempi del processo. Queste persone hanno il diritto di essere giudicate nel più breve tempo possibile ed è impensabile che, per un *deficit* dello Stato, debbano pagare i cittadini. In uno Stato civile e democratico ciò non dovrebbe mai accadere, mai, per nessun motivo motivo ed è la nostra Carta costituzionale, sono i principi fondanti del nostro sistema processuale a imporcelo. Questo Governo - è innegabile si è ritrovato a dover fronteggiare una situazione difficile e complicata ed apprezzabile è il tentativo, seppur a tratti maldestro, di porre un argine a quanto di assurdo è stato fatto, o non è stato fatto, negli anni passati. Non può sottacersi, però, come tutto ciò che verrà fatto da adesso in poi sarà - questo sì - di responsabilità di chi governa. Voi oggi avete la possibilità di mettere finalmente la parola fine a una delle pagine più becere

Voi oggi avete la possibilità di mettere finalmente la parola fine a una delle pagine più becere e vergognose dell'edilizia giudiziaria nel nostro Paese, dando risposte certe e definitive e avendo il coraggio di scegliere al di là degli interessi dei singoli. Tutto questo tenendo bene a mente, però, i valori della nostra Costituzione, infranti di fronte alla scelta di sospendere la prescrizione e ascoltando le grida, le preoccupazioni e i suggerimenti dell'avvocatura barese, soprattutto dei più giovani, che, avvicinatisi a una così nobile e antica professione, si trovano oggi nell'impossibilità di lavorare e, nel contempo, sottoposti regolarmente agli obblighi contributivi e fiscali.

il fascismo cadeva a seguito della votazione da parte del Gran consiglio dell'ordine del giorno presentato da Dino Grandi. Un fatto storico, apparentemente lontano, apparentemente lontano, ma che invece parla ancora oggi alla nostra vita democratica: fu quella la data che segnò il primo passo verso il recupero del percorso democratico per il nostro Paese. Sembrava che finalmente fosse finito tutto, il fascismo, la guerra. Quel giorno molti italiani scesero in piazza per festeggiare. Invece il Paese doveva ancora vivere molti mesi cupi di guerra civile e di scontro con il nazifascismo. Ci fu la grande campagna partigiana, che portò al 25 aprile del 1945 e alla definitiva liberazione del nostro Paese. fondante del percorso per la democrazia nel nostro Paese. Benito Mussolini quando divenne capo del Governo fece alla Camera dei deputati alcune affermazioni pesantissime; disse: «potevo fare di questa Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli; potevo sprangare il Parlamento e costruire un Governo esclusivamente di fascisti. Potevo; ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto». Sappiamo come proseguì la vicenda del nostro Paese. In questi giorni - e lo dico davvero senza nessun intento di associare storicamente i due passaggi - c'è stato chi ha detto il Parlamento potrebbe anche essere abolito un domani. Allora io dico che dobbiamo fare molta attenzione, ricordando anche il percorso storico del nostro Paese, perché la democrazia rappresentativa forse necessita forse necessita di alcune ristrutturazioni e di alcuni aggiustamenti, ma un conto è aggiustare un processo e un percorso che nascono da una storia importante, altra cosa è pensare di abolirlo In quest'Aula, sopra la Presidenza, c'è un cartello che ci ricorda come la Repubblica italiana sia stata proclamata a presidio di pubbliche libertà e a certezza del progresso civile. La data del 25 aprile, la data della caduta del fascismo, continui a dirci che quella è la strada che dobbiamo proseguire, aggiustando, se necessario, il percorso della democrazia. Accanto a quell'avvenimento ci fu da parte della famiglia Cervi un'iniziativa incredibile: l'offerta di una pastasciutta in piazza per festeggiare la caduta del fascismo, nella consapevolezza o, meglio, nella speranza, che davvero fascismo e guerra fossero terminati. Quell'iniziativa, da circa vent'anni, viene ripetuta non solo nella sede dell'Istituto Cervi, ma in molte piazze e città italiane. Accadrà questa sera in tante parti d'Italia che molti cittadini si riuniranno per rivivere lo spirito dell'antifascismo e della Resistenza. Credo che sia bello poterlo ricordare in quest'Aula e in questa giornata speciale, a settantacinque anni dalla caduta del fascismo.

è di poche ore fa la notizia di un incendio, l'ennesimo, ancora in corso tra l'altro, che ha investito un sito industriale di stoccaggio e trattamento dei rifiuti nella zona industriale di Pascarola, in provincia di Napoli. Le immagini che sono state diffuse sono impressionanti; c'è una nube nera altissima che sta ricoprendo i Comuni di Caivano, di Orta di Atella, di Crispano, che è visibile a chilometri di distanza. È una nuova sciagura ecologica, l'ennesima, a cavallo tra le province di Napoli e Caserta, in una delle zone urbane più densamente popolate della Campania e che ricade in quel territorio oramai tristemente conosciuto come Terra dei Fuochi. Le istituzioni sono state allertate e sul posto sono intervenute le forze di polizia e i Vigili del fuoco, eroi silenziosi in una guerra impari che dura ormai da troppi anni e ai quali va tutto il nostro sostegno e il nostro ringraziamento. Si tratta dell'ennesimo rogo che in poco tempo ha investito anche diversi siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti solidi urbani e questo pone un grosso interrogativo anche rispetto alle misure di sicurezza impiegate dagli operatori autorizzati al trattamento dei rifiuti in Campania. Ciò che è preoccupante, però, è che dai primi riscontri l'incendio di oggi, ancora una volta, sembrerebbe avere un'origine dolosa. Le autorità competenti sono già al lavoro per fare luce su questo aspetto che, se confermato, assumerebbe un carattere di una gravità inaudita a riprova, qualora ancora ce ne fosse bisogno, dell'esistenza di un disegno criminoso ormai consolidato che investe l'intero comparto di trattamento e smaltimento dei rifiuti in Campania. È un disegno criminoso che interessa direttamente la salute di un popolo campano sempre più esasperato, sempre più stanco. Non è più rinviabile l'introduzione di misure di sicurezza specifiche, stringenti e anche, perché no, si potrebbe pensare alla militarizzazione di quei siti di stoccaggio che insistono in quest'area ad alto rischio di azioni criminose e scellerate, a tutela sia dell'integrità dei siti stessi,